L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Viceversa, voglio essere ulteriormente collaborativo e raccontarvi come vedrei io il bilancio. Lo vedrei scritto su una lavagna, ma siccome adesso siamo arrivati alle *slide* e a ben altri mezzi, accetto la *slide*

So che gli economisti di una volta dicevano che uno starnuto a Hong Kong era una polmonite a New York, per cui una notizia in economia data male può causare variazioni - di miliardi, nel nostro caso - tali per cui siamo poi costretti a correre dietro a tagli

per le pensioni, 110 per la sanità, gli stipendi, la manutenzione degli edifici e spese fisse varie, ci sono 5-10 miliardi discrezionali,

nelle promesse elettorali, nelle scelte discrezionali del Governo e nella politica). In questi importi dovrebbero rientrare anche gli investimenti, che temo siano e saranno pochi, sia per le procedure, sia perché si confida

per 14 miliardi, che sono spese correnti e soldi che dall'Italia vanno all'Europa. Ai tempi in cui essa fu istituita, questi fondi provenivano dall'IVA, oggi provengono in generale dal bilancio. Ne riprendiamo 12 circa, ma non sempre, perché non siamo capaci di usare i fondi europei, dato che ci mancano i co-finanziamenti, soprattutto al Sud. Questi sono i fatti. Dove vanno i soldi che non vengono ripresi in corso d'anno? A residuo? E comunque ci sono 2 miliardi che costituiscono la perequazione a Est dell'Europa e le spese faraoniche della stessa. Poi l'Europa ci mette le norme sull'etichettatura dei prodotti, soprattutto quelli alimentari e dobbiamo fare la guerra. Ci dice, ancora, che sui citofoni non dobbiamo scrivere il nome. Queste sono le misure che dobbiamo contestare all'Europa. Qui dentro, però, il problema è il debito pubblico. Io vorrei che si facesse un'apposita discussione sul debito pubblico per cercare di ridurlo, con la proposta di Savona, Panerai e altri della costituzione di una società con patrimonio immobiliare pubblico, vendita delle quote

del sottosegretario Giorgetti e di altri, e gliene do pubblicamente atto. Altre norme riguardano gli avanzi di amministrazione, il bilancio consolidato per i piccoli Comuni, la contabilità economico-patrimoniale, di cui spero sia stata salvata l'abolizione, e la soglia degli appalti

sapere che si governa per tutti, non soltanto per quelli che si presume abbiano votato. Si governa per tutti, perché questo è il passato, il presente e il futuro.

Signor Presidente, anch'io, come diversi parlamentari ieri sera, devo stigmatizzare la condotta del Governo nei confronti del Parlamento sulla legge di bilancio. Si è trattato, lo dico con serena gravità, di un vero e proprio atto di disprezzo del Parlamento. Il senso di responsabilità del Parlamento permetterà forse di evitare l'esercizio provvisorio,

Ad una vera mancanza di tempo perché il Governo è entrato in carica solo da poche settimane? Ad un'improvvisa crisi che ha stravolto lo scenario economico-finanziario internazionale? No, non vi è alcuna circostanza attenuante di questo tipo.

Senatore, pensavo che, senza averla nominata, avesse compreso a chi era indirizzato il richiamo. Non mi costringa a richiamarla nominalmente.

che forse è l'unico elemento che le due forze politiche della maggioranza hanno veramente in comune. Aggiungo il disprezzo dei numeri, spesso derubricati a numerini; è anche questo un aspetto della non presa d'atto della realtà, salvo che poi i numerini vengono resi ancora più numerini quando può essere utile usare, per la prima volta nella storia delle relazioni tra l'Unione europea e uno Stato membro, due cifre decimali. Un Governo, che con orgoglio si considera sovranista e populista rifiutandosi per mesi di avere un dialogo serio con una realtà considerata ostile e da travolgere, l'Unione europea, ha finito per capitolare davanti agli eurocrati. Ha rinviato di giorni e giorni e poi ancora di un'ora due giorni fa (dalle ore 12 alle ore 13) la presentazione della manovra in Senato, perché non arrivava la lettera di nulla osta da Bruxelles. Il Governo sovranista ha ottenuto il risultato di cedere all'Europa in modo maldestro una quota rilevante della sovranità nazionale italiana sottraendola a chi? Il Governo populista ha tolto sovranità al Parlamento che, come ha ricordato l'altro ieri il presidente Mattarella, è interprete ed espressione della sovranità popolare. Quindi, c'è stata una perdita netta di

manovra in condizioni particolarmente favorevoli. Guardando almeno gli ultimi dieci anni, nessun Governo italiano si è trovato a dover essere confrontato con un'economia ricevuta dal passato non certo florida, ma che, superata una grave crisi finanziaria e una severa recessione, dà o dava - dovremmo forse dire - segni di ripresa. I mercati finanziari e la politica monetaria non erano mai stati così favorevoli. Ricordiamo tutti il *quantitative easing*. easing*. Va anche detto che le condizioni politiche della maggioranza rispetto alla debolezza numerica e - mi si permetta di dire - di idee delle opposizioni avrebbero potuto favorire una rigorosissima azione di Governo.

Vi ricorderete cosa rischiava di voler dire il contagio della Grecia qualche anno fa. Questa volta siamo stati così fortunati da subire per dono di Dio il contagio, nel senso dell'allargamento, dovuto all'azione dei *gilet* gialli in Francia e alla duplice circostanza che il commissario Moscovici è molto politico e molto francese. Credo che senza queste circostanze, come si legge anche in qualche giornale di oggi, quella coalizione di Stati membri del Nord falchi e cattivi non avrebbe consentito alla Commissione di risparmiare l'apertura della procedura di infrazione verso l'Italia. L'abbiamo effettivamente scampata bella. Io vorrei soffermarmi per un attimo su come mai all'ultimo minuto il Governo italiano sia riuscito effettivamente a riprendere la situazione in mano. Secondo me, bisogna capire come prima si sia verificato un tale degrado del quadro di negoziato con l'Europa e come poi si sia potuto rimediare in pochi giorni. Tutti abbiamo esperienza di funzionamento di istituzioni, di aziende e di politica. Di solito, quando un comportamento va storto, quando una *performance* è cattiva una parte della ragione risiede nella nella cattiva struttura delle istituzioni oppure nel fatto che le istituzioni non vengono fatte funzionare come sarebbe prescritto. Bene. Io credo che abbiamo avuto grandissimi problemi, rimediati all'ultimo minuto ma con danni effettivi per il Paese perché per mesi e mesi la politica economica e la politica europea sono state condotte, nelle loro manifestazioni più visibili, da Ministri non competenti e non responsabili. Per la politica economica ha avuto forse anche eccessiva attenzione - ma è stato citato da tutti - l'atto del balcone del vice presidente Di Maio. Dopo avere sconfitto il competente Ministro dell'economia, l'ha fatto sapere al mondo. Ma non vorrei che si sottovalutasse il contributo dato in questo senso, cioè alla creazione di un pessimo ambiente negoziale con l'Europa, dal vice presidente Salvini che non ha avuto a disposizione in modo puntuale e trionfale un balcone, ma infiniti microfoni collocati in stadi, birrerie, sagre e altrove, dalle quali ha formulato, con martellante puntualità, la politica estera e la politica europea dell'Italia. Nei giornali internazionali la politica estera ed europea dell'Italia era quella dichiarata, giorno per giorno, dal Ministro degli interni. Ebbene, se voi ci fate caso, le cose si sono un po' raddrizzate quando è successo nel funzionamento del Governo quello che colpevolmente prima non era stato fatto succedere dal Presidente del Consiglio dei ministri: lui ha cominciato a guidare il Governo, sono riapparsi per la politica economica il ministro Tria e per la politica estera il ministro Moavero Milanesi e le cose sono andate meglio. meglio. Io spero sempre nella stabilità dei governi, che in genere migliorano via via che imparano, purché non rifiutino il confronto con la realtà per la stabilità e l'efficacia del Governo mi auguro che il Presidente del Consiglio sappia fare tesoro di questa esperienza. Aggiungo un paio di ultime considerazioni: ho rilevato, al momento del primo dibattito sulla fiducia, che questo Governo e questa maggioranza sono costituiti dagli unici due partiti che hanno avuto un travolgente successo elettorale che hanno costruito, in gran parte, sulla base di una narrazione falsa, di una storia alla quale hanno partecipato solo per distruggere, cioè sono stati i due unici partiti che, a differenza del PD, di Forza Italia e dei partiti di centro che c'erano allora, non si sono assunti alcuna responsabilità nel far uscire l'Italia dalla crisi del 2011-2012. Ebbene, hanno costruito una narrazione che adesso, se vogliono governare, devono smontare pezzo per pezzo. Ma io assicuro ai colleghi della Lega e dei 5 Stelle che mai dirò che con la ritirata poco elegante che ci hanno fatto vedere in questi giorni siano stati servi dei poteri forti, del capitalismo internazionale, inginocchiati di fronte alla Commissione europea e altre delizie con le quali hanno caratterizzato il loro contributo critico alla vita politica italiana degli ultimi sei o sette anni. Infine, a proposito sì, nelle intenzioni devo dire che a me piaceva moltissimo l'idea che fosse una manovra del popolo, ma sapete "del" in italiano può denotare soggetto o oggetto. È nata come manovra del popolo, fatta dal popolo nell'interesse del popolo, ma è diventata moltissimo alla fine - e mi dispiace - un atto di manovra sul popolo nel quale sono state fatte penetrare idee di vittoria, di benessere futuro incrementato, di

adesso converrebbe, contenuto il pur giustificato, in parte, giubilo per aver evitato la procedura di infrazione, concentrarci sulle prossime tappe. Le leggiamo bene nei giornali oggi e, in parte, le abbiamo costruite noi: una sorta di mercato dei tappeti, anzi tappeti volanti, sotto i quali c'è moltissima polvere in forma di IVA per i prossimi anni. Quindi, grandissima attenzione, perché non siamo ancora ad una Italia liberata da un'Europa che esiste e che esercita la sua sorveglianza perché tutti i Paesi le hanno chiesto di esercitarla.

perché di testi ne abbiamo avuti molti, ma mai quello sul quale lavorare definitivamente. L'*iter* di questa manovra è l'emblema della approssimazione dimostrata quasi quotidianamente questi primi sei mesi di Governo. Balletti penosi, cifre, misure, emendamenti, previsioni surreali di crescita, attacchi all'Europa, meste retromarce e autosmentite come quella, ad esempio, sulla tassa sulle auto più inquinanti. Per giorni, un evidente tentativo di prendere tempo perché, ce ne siamo accorti, ci si è dovuti limitare a discutere di misure minori, sostanzialmente mance e mancette distribuite senza

non sono stati finora chiariti in modo definitivo. Questo in particolare per quanto riguarda le vostre misure principali, che sono la quota 100 e anche il reddito di cittadinanza, che non sappiamo ancora come verrà erogato, che cosa ci si farà e cosa vi è scritto dentro, a parte qualche tessera che forse stanno stampando. Ci è stato detto che in Senato sarebbero arrivate le vere modifiche. Ebbene, noi siamo ancora qui ad aspettare le modifiche. A parte la relazione del presidente Conte, che ci ha detto che vi saranno ulteriori tagli, quindi, noi stiamo aspettando per sapere dove saranno effettuati questi tagli. Alla fine, la legge di bilancio che verrà fuori da quest'Aula si limiterà solamente a sollevare molto fumo e un po' di assistenzialismo, senza promuovere la crescita, senza diminuire le tasse e senza mettere in cantiere investimenti di cui il Paese avrebbe bisogno. Si tagliano fondi anche all'università perché, con il blocco del *turnover* da novembre del prossimo anno, non abbiamo fatto altro che bloccare i fondi all'università. Inoltre, i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che non avete voluto audire in Commissione, già allora ci dicevano che ci sono sei miliardi di euro in più e che poi il prossimo congelamento con la manovra sull'IVA porterà, nel 2020 e nel 2021, ulteriori tasse sulla testa dei cittadini. Sarebbe stato opportuno proseguire sulla strada delle riforme avviate nella precedente legislatura e, di fatto, voi lo avete fatto. Infatti, con il Rei, il reddito di inclusione, avete comunque recuperato e avete già inserito in questa manovra norme che possono mantenerlo in vita fintanto fintanto che non verrà approvata. Questo perché vi siete accorti che questo famoso reddito di cittadinanza non ha ancora né testa né coda. Sarebbe stato opportuno non sfidarla l'Europa. Ma tant'è, voi l'avete sfidata dicendo sempre: "Me ne frego" e "Noi andiamo avanti", per poi ritornare a dire che è meglio che stiamo

nessuna programmazione di sistema, solo annunci a *spot*. Il Fondo sanitario nazionale è rimasto uguale a quello programmato dai Governi precedenti, non si è spostato di una virgola. Alla faccia dell'elenco del *premier* Di Maio, che dice: «Fatto!».

liste d'attesa sono stati messi 50 milioni di euro e aggiunti altri 150, ma tutto per l'implementazione della cosiddetta «rete tecnologica». Non capisco: bisognava assumere i medici per fare le visite, non avere un'informatizzazione migliore. Per non parlare, poi, del superticket, altro proclama importantissimo:

annunciando un altro sciopero; uno è già stato fatto e ne stanno preparando un altro. Ci sono 120.000 dirigenti che non sono mai stati incontrati dalla Ministra. Inconcepibile, poi, quello che sta succedendo in sanità: azzerato il Consiglio superiore di sanità con una lettera. Si tratta di gente che ha lavorato per quattro anni gratuitamente a livello scientifico: cancellati con una lettera. Qui si procede a raccomandate per cancellare le eccellenze italiane.

con il tetto per l'assunzione del personale in sanità: anche su questo, proclami, ma di fatto non si sa niente. Chissà se sarà nel prossimo maxiemendamento, che arriva oggi pomeriggio, perché la Ministra, insieme a Garavaglia, aveva detto «faremo, faremo», però non abbiamo ancora visto niente di definitivo. Desta, poi, una preoccupazione - che credo che le donne qui presenti debbano sentire propria - il fatto di aver riconosciuto alla lavoratrici la facoltà di estendere il lavoro dopo il parto per cinque mesi, in deroga alla legge vigente, che prevede che stiano a casa i due mesi prima e i tre mesi dopo. Nonostante si tratti di un'operazione volontaria, tale norma espone ovviamente le donne alla possibilità di pressioni e di condizionamenti da parte dei datori di lavoro, che rischiano di mettere in pericolo la salute della donna stessa e del nascituro. Ricordate che non tutte le donne lavorano in ufficio; ci sono tante donne che lavorano e fanno lavori faticosi. Signor Presidente, non possiamo negare di essere fortemente preoccupati. Vi abbiamo implorato, nell'interesse del Paese, di riscrivere la manovra, di accogliere le nostre proposte. Vi abbiamo offerto collaborazione, ma, devo dire, da parte vostra vi è stato un finto ascolto: non c'è stato nessun dialogo, né alcuna disponibilità vera. manovra del popolo, ma della recessione, portata avanti dal Governo non del cambiamento ma del fallimento di un Paese che non se lo merita. Perché l'Italia non si merita questa manovra.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, se guardo a quanto è accaduto in quest'ultimo periodo, mi rendo conto che l'Italia sembra essere stata portata a una condizione borsistica. In pratica, il Paese ha come priorità principale la verifica delle quotazioni.

praticamente, sarebbe bastato qualche punto percentuale in più tra entrate e uscite e saremmo stati davanti non più ad uno Stato, ma ad una banca, che però si trova in una condizione prefallimentare, se non già in liquidazione. A me sembra che questo sia un aspetto che merita molta attenzione, come meritano ancora più attenzione le dinamiche che hanno portato il Paese in questa particolare condizione. Ovviamente ora tocca a noi governare il Paese, mentre in precedenza è toccato ad altri. Noi, però, ci assumiamo la responsabilità di governare il Paese e di farlo bene. Mi sembra che si sia persa l'attenzione sull'elemento principale per cui siamo qui, che è rappresentato dai cittadini e non certo dai mercati finanziari. Vorrei evidenziare alcuni aspetti che più volte sono stati richiamati in questi giorni. Si tende sempre a parlare della parte di competenza del bilancio - uso un tecnicismo - e nello specifico delle entrate e delle uscite. Non ho mai sentito parlare, però, o almeno non con la frequenza che meriterebbe, del fatto che lo Stato non è più in grado di fare fronte alle spese correnti con le entrate tributarie e questo è un problema gravissimo *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché significa che non c'è la sostenibilità finanziaria naturale, da tempo, di un organismo complesso quale è il nostro Paese. Perché è accaduto tutto ciò? Questo aspetto ha certamente incattivito anche il sistema tributario italiano, che è datato - ecco perché abbiamo parlato di riappacificazione fiscale con i cittadini - che negli anni è stato pensato per aggredire i contribuenti, soprattutto quelli più ricchi, e che non si è adattato tempi a ad un mondo che ormai da decenni. La globalizzazione non si è certo realizzata ieri mattina: sono anni che il nostro Paese è inserito in un mercato globale, dove anche gli altri Paesi hanno vissuto - penso ad esempio alla crisi dei mutui *subprime* - ma hanno avuto una migliore capacità di uscirne rispetto a noi. dunque, è accaduto tutto questo? Perché abbiamo - ad esempio - dei differenziali positivi? Torno ancora una volta a un tecnicismo: parliamo di legge di bilancio e, dunque, i tecnicismi sono necessari o almeno apparentemente positivi, se vogliamo vedere piccoli particolari del bilancio, che poi però si scontrano con parametri finanziari profondamente negativi, se vogliamo analizzare altre sezioni molto importanti del bilancio. Come ho detto più volte, anche in altre occasioni, continuo a chiedere ancora: chiedere ancora: se quei crediti benedetti presenti nello stato patrimoniale del bilancio statale, che sono i ruoli che non vengono riscossi - si tratta di 900 miliardi di euro restano lì e non vengono riscossi, allora i differenziali finanziari del bilancio dello Stato si moltiplicheranno in negativo in maniera esponenziale? Che effetto avranno sul debito pubblico? Quindi, quandanche avessimo un minimo miglioramento del debito pubblico, la situazione finanziaria rimarrebbe comunque tendenzialmente negativa ed è tale da anni, come accade ancora e non

cui aggiungerei anche una quarta pagina, contenente i *report* della Banca l'Italia sul debito pubblico. A questo punto avremmo dato agli italiani la rappresentazione certa di una situazione finanziaria sistematicamente deficitaria e negativa, quella con la quale oggi ci stiamo confrontando. È quello il parametro del successo mancato delle politiche economiche adottate negli ultimi anni, quella che avete portato avanti voi, che oggi pensate di essere maestri della nostra politica economica.

il problema di prima - lo Stato deve accendere prestiti, allora capisco che quei prestiti serviranno a restituire altri prestiti. Ecco perché lo *spread* spaventa: diciamolo ad alta voce. Lo *spread* spaventa perché, negli ultimi vent'anni, l'Italia è stata fortemente indebolita dal punto di vista patrimoniale e in modo particolare da quello finanziario, con una crescita del debito spaventosa, minimamente contenuta solo negli ultimi anni, in conseguenza di regole europee che vanno bene solo per un Paese che non ha però un debito pubblico come quello italiano. italiano. Bisognerebbe, quindi, in tanti chiedere scusa agli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ma chi ha ridotto il Paese in queste condizioni? Chi ha aumentato il debito pubblico? Ora per quale motivo per ripianare debito pubblico, con miglioramenti millesimali, si mette in discussione lo Stato sociale a tutti i livelli, oltre che la sopravvivenza stessa dei cittadini e delle imprese? Stiamo dunque lavorando con un atto di coraggio ed è più che giustificata la confusione in cui ci troviamo, perché - da un lato - abbiamo ereditato una condizione di grande precarietà nazionale a tutti i livelli sociali, dalla sanità alle pensioni, dalle scuole ai disoccupati, alle casalinghe e alle imprese, mentre - dall'altro lato - siamo chiamati a fare fronte e a muoverci all'interno di regole europee che sono state previste per Paesi sicuramente meno gravati dal debito pubblico rispetto all'Italia. Ma chi lo ha creato questo debito pubblico? M5S)*. Quando leggo che il debito pubblico è migliorato e dovrei esserne felice, mi chiedo: a quale prezzo? Nell'ultimo rendiconto di gestione, per il quale sono stato relatore, ho trovato passività finanziarie solo in aumento. Abbiamo un debito pubblico che è dopato anche quando migliora da un sistema finanziario che finisce con istigare il sistema fiscale a essere iperaggressivo nei confronti dei cittadini e, siccome non riesce a intercettare i contribuenti più importanti e più ricchi, si accanisce sui restanti, la massa, la quale non è in grado a volte di pagare. In tutto questo, perché abbiamo residui attivi, che sono soldi che abbiamo tutto il diritto di recuperare, che non vengono incassati? I ruoli aumentano sempre più di numero e vanno ad aggiungersi a un'evasione fiscale che si aggira intorno ai 210 miliardi di euro. Ecco allora che quelli che vengono intercettati vengono anche aggrediti dal fisco. aggrediti dal fisco. Mi rendo conto che il sistema è malato, ma, da semplice ignaro, direi che tutto ciò che c'è di sbagliato è stato fatto in precedenza e viene testimoniato in maniera inequivocabile non dalle mie parole, ma da due elementi più che negativi: il debito pubblico e le passività finanziarie, aggravate dall'incapacità dello Stato di riscuotere i tributi. tributi. È stato fatto bene? No, non è stato fatto bene finora. Allora è giusto andare a rivedere il sistema Paese nel suo complesso ed è giusto andare a recuperare il rapporto con l'Europa, che ha delle regole certamente molto stringenti, ma che bisogna rispettare nel momento in cui ne facciamo e continueremo a farne parte, anche se l'Europa non si fida dell'Italia

dal rendiconto di gestione dello Stato 2017 e del *report* della Banca d'Italia, che hanno evidenziato in maniera inequivocabile il fallimento delle vostre politiche economica finora attuate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ora tocca a noi provare altro e, a dispetto dei dubbi del caso, l'Italia ci chiede di cambiare rotta e noi la stiamo cambiando.

Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Presutto che siamo a dicembre del 2018

senatore Presutto, si stanno congratulando tutti, ma il discorso che ha fatto poteva farlo - e sicuramente lo avete fatto lei o alcuni suoi colleghi - uno, due o tre anni fa e non a fronte della manovra economica che voi avete realizzato in questo Parlamento e che aggrava tutto quello che lei ha detto, peggiorando la situazione e il rapporto con l'Europa. E ciò avviene non solo perché siamo stati due mesi

che nella nuova formulazione diventa solo una rete di sicurezza per le banche dei Paesi del Nord Europa. Collega Presutto, ha capito? Avete accettato una riforma del fondo salva Stati, che è una rete di protezione solo per le banche del Nord Europa. avvenuto nel Consiglio europeo di pochi giorni fa e non tre, quattro o cinque anni fa; è accaduto nel vostro Governo. Nello stesso Consiglio europeo avete accettato una riforma che rende meno appetibili i titoli pubblici italiani. Avete capito? Avete barattato questa manovrina del 2 per cento svendendo i titoli pubblici italiani. Avete accettato nello stesso Consiglio europeo un nuovo bilancio della zona euro che di fatto finanzierà solo i Paesi che sono in regola con i vincoli europei e, quindi, non l'Italia. Avete rinunciato, sempre allo stesso Consiglio Europeo, alla richiesta di garanzia europea sui depositi, che era già prevista dall'Unione bancaria: avete svenduto non solo la manovra economica, ma lo stesso futuro dell'Italia, pur di far passare qualcosa che sia una manovra di sapore elettorale per le elezioni di aprile e maggio. Questo è il conto che dovete portare agli italiani, peraltro un conto di cui gli italiani si stanno accorgendo. Chiedetevi per per quale motivo, un giorno dopo l'altro, abbiamo avuto intorno al Parlamento prima il blocco dei noleggiatori, il giorno dopo il blocco selvaggio dei tassisti e il giorno dopo ancora il blocco dei bus turistici. Non sono i ricchi che stanno facendo i blocchi,

e sono bruciate da poveri proletari, malgrado voi abbiate realizzato una manovra che è un esproprio proletario. È un esproprio proletario nei confronti del Parlamento, di questa istituzione borghese che va espropriata nelle sue prerogative al punto tale che ancora non abbiamo la manovra di bilancio. Ma è un esproprio proletario nei confronti dei ceti produttivi, dei lavoratori e di chi in questo Paese fa economia e benessere

C'era un cappio scorsoio sui beni e sui consumi degli italiani e quel cappio voi non l'avete levato agli italiani, ma lo avete aggravato. Lo stesso vale per le imprese: non c'è una misura a sostegno delle imprese, anzi vengono tolti soldi in più; oltre a quelli che avete tolto alla Camera, se vedete la tabella del vice ministro Di Maio, leggerete soltanto più tasse, più entrate fiscali e, quindi, più pressione fiscale per le imprese e per chi lavora. Faremo un manifesto dopo questa legge finanziaria che elencherà

ci sarà scritto: «Taci e paga, somaro del Nord». Questa legge finanziaria, la prima fatta compiutamente dai 5 Stelle e dalla Lega, è un esproprio proletario, ma non in favore dei proletari.

ma solo qualcosa - in campagna elettorale. Questa è una non manovra proletaria, ma elettorale. Non è una manovra espansiva, ma è una manovra recessiva. Non è una manovra per il popolo, ma è una manovra contro il popolo. Questa è una manovra che avete subìto dall'Unione europea per quanto riguarda i parametri, che avete scritto, con una sorta di analfabetismo economico, sulla base di un rancore qual è quello che voi avete nei confronti di chi ha prodotto ricchezza in questo Paese,

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, vorrei anzitutto tranquillizzare il nominato senatore a vita Mario Monti che noi non possiamo prendere lezioni da chi ha messo in ginocchio economicamente il nostro Paese con un Governo mai votato dagli italiani - come d'altronde lo è anche lui - e imposto proprio da quei poteri occulti che ogni giorno ostacolano l'azione di questo Governo del cambiamento, che - lo dico in modo chiaro - non si inchinerà mai più a chi non ha a cuore il bene di tutti gli italiani. Prima gli italiani, sempre! Intervengo, signor Presidente, su un settore specifico che è stato richiamato anche ieri, il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare, che vale 140 miliardi di euro per il nostro Paese - lo ricordo in quest'Aula

una su tutte, che è stata messa in discussione e rappresenta il ricambio generazionale, una nuova opportunità di lavoro: l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli a partire dal 2019, 2020 e 2021. Quelle famiglie potranno anche richiedere un mutuo, fino a 200.000 euro a tasso zero, per costruire l'abitazione vicino ai terreni dove sono insediate. Proprio questo Governo, che sembra non far nulla per il settore, anche e soprattutto per le zone di montagna ha finanziato il Fondo nazionale per la montagna con 10 milioni di euro l'anno 2019, 2020 e 2021. C'è poi la promozione dei nostri prodotti, di cui parliamo sempre. Abbiamo approvato un ordine del giorno in quest'Aula, con un punto specifico che chiedeva al Governo di promuovere di più il *made in Italy* nel mondo; è stato finanziato con 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020. Signor Presidente, le chiedo la cortesia di darmi qualche minuto in più. PRESIDENTE. Qualche minuto in più è impossibile; al massimo le posso concedere 30-40 secondi. di segnalare l'importanza di una misura che è stata sottoscritta da tutti i Gruppi presenti in quest'Aula e che, se approvata nella legge di bilancio, andrà a definire una carenza normativa fiscale relativa alla raccolta occasionale di prodotti selvatici (funghi, piccoli frutti, tartufi e erbe officinali). La stima è che la popolazione interessata dalla proposta possa arrivare addirittura a due milioni e mezzo di italiani; di queste persone, circa un milione utilizzerà la norma proposta, ovvero le persone che dalla raccolta ricavano più del 10 per cento del loro reddito familiare. Segnalo che c'è una legge, la legge n. 122 del 7 luglio 2016, che è stata devastante per il settore dei tartufi, con una perdita dell'85 per cento dell'approvvigionamento di prodotto nazionale e del 60 per cento a livello europeo del prodotto italiano. Noi vogliamo mettere fine a questo scempio pericoloso, soprattutto perché c'è un vuoto normativo; vogliamo difendere il nostro *made in Italy*. Il settore va messo nelle condizioni di poter operare con la massima trasparenza;

Signor Presidente, onorevoli colleghi, almeno per ora la procedura d'infrazione europea sembra sventata, meno male, ma a che prezzo? Il Parlamento è stato totalmente esautorato: è la prima volta che il 21 dicembre qui in Parlamento non si conoscono ancora i dettagli della manovra

per costruire scuole, ospedali, autostrade. Ci siamo fatti compatire a livello internazionale, signor Presidente, salvo poi andare a pietire un compromesso al ribasso col cappello in mano. Il risultato è che la manovra, per la prima volta nella storia del Paese, è stata scritta direttamente da Bruxelles. Altro che Governo sovranista! Al dunque, quando si tratta di difendere l'Italia, l'Esecutivo si fa dettare i conti in casa propria, tra l'altro sminuendo totalmente il ruolo del Parlamento e tradendo anche quelle promesse populistiche che ci hanno portato all'attuale drammatica situazione. Questa manovra disattende e tradisce totalmente le promesse fatte dal Governo giallo-verde. Innanzitutto non smonta la legge Fornero sulle pensioni, anzi prevede una stangata di 2,5 miliardi sulle pensioni a partire da quelle da 1.500 euro, che non mi pare siano pensioni definite d'oro;

e torna a congelare lo sblocco del *turnover;* quello sblocco del *turnover* che noi avevamo deliberato, ma adesso per le assunzioni nella pubblica amministrazione dovremo aspettare ancora un anno. anno. Soprattutto poi questa manovra non investe né in crescita né in sviluppo; in parte distribuisce in modo diverso le risorse che avevamo stanziato con i nostri Governi a ma non prevede misure a favore del lavoro né dell'impresa; cancella tutta una serie di agevolazioni fiscali che avevamo introdotto. La questione è la seguente: se non si produce ricchezza, chi paga? chi paga? Infatti, aumenta consistentemente il debito pubblico, andando a gravare pesantemente sulle giovani generazioni. La manovra pone inoltre pericolose ipoteche sul futuro di questo Paese, non soltanto prevedendo un incremento fortissimo dell'IVA a partire dal 2022;

determinando quindi un danno forte, non soltanto per le nostre comunità nel mondo, ma per l'intero sistema Paese. Anche sulle questioni della Difesa la situazione non è migliore. Per come è scritto, il disegno di legge di bilancio non dà alcuna chiarezza su dove vadano a incidere i tagli previsti nel citato Al di là di qualche discordante dichiarazione dei singoli Ministri, le uniche informazioni che abbiamo sono quelle ricavate da un comunicato stampa dell'Esecutivo, reso pubblico il 15 ottobre scorso, sui contenuti del disegno di legge di bilancio. Nell'unico passaggio in cui si parla di Difesa si afferma che si prevede una riduzione delle spese militari pari ai fondi necessari per la riforma dei centri per l'impiego. inutile dire che non può esserci un approccio peggiore nei confronti del comparto della Difesa, un settore che più di ogni altro all'interno della pubblica amministrazione necessita di una programmazione a lungo termine e di una ragionevole certezza delle risorse e degli investimenti. Un atteggiamento simile, dunque, non può che denotare scarsa considerazione e consapevolezza delle esigenze di un comparto che ricopre, invece, un ruolo delicatissimo e decisivo per il Paese non solo per la sicurezza interna, ma anche per la dimensione internazionale e lo sviluppo economico dell'Italia.

denotano la mancanza di un chiaro indirizzo strategico e la totale assenza di visione politica in ambito di difesa. Per di più, questi tagli creano sul nostro sistema di sicurezza, sull'intero comparto tecnologico e industriale e sulla credibilità internazionale del nostro Paese una forte incertezza, con gravi effetti a livello operativo, industriale e internazionale.

è avvilente e offensivo non soltanto per gli uomini delle nostra Forze armate, ma anche per la stessa città di Roma. Le donne e gli uomini del nostro Esercito hanno compiti ben diversi dall'essere impiegati come tappa buchi, per svolgere riparazioni che dovrebbero rientrare nell'ordinaria amministrazione della Giunta. Per di più, si tratta di una Giunta che solo pochi mesi fa ha detto no alle Olimpiadi

Insomma, signor Presidente, se questa è la manovra del cambiamento, povera Italia! Poveri noi!

Come promesso, supereremo la legge Fornero e introdurremo quota 100. Abbiamo investito tante risorse nella sanità e quasi 600 milioni di risorse aggiuntive nel sociale. tante misure per scuola, università e ricerca, nonché il fondo di 525 milioni, per tre anni, per ristorare i risparmiatori truffati. per le imprese, di cui la Lega ha profonda cultura; abbiamo raddoppiato la deducibilità dell'IMU dei capannoni ed esteso il regime forfettario. Stiamo parlando di 1,5 milioni di partite IVA, che, con ricavi inferiori a 65.000 euro,

per le plastiche e bioplastiche monouso - ne parlerà dopo il collega Briziarelli - grazie a una norma introdotta dalla Lega, viene salvato un comparto di decine di imprese italiane, con 3.000 dipendenti e un fatturato di oltre un miliardo, che rischiava di chiudere. *(Applausi

sono stati introdotti spazi finanziari per i Comuni, che potranno così utilizzare gli avanzi di amministrazione per fare investimenti necessari alla ricostruzione.

che questo Governo e la Lega hanno a cuore le comunità terremotate, alle quali non mancherà mai l'azione di sostegno. *(Applausi dai di prorogare la vita utile degli impianti di risalita dei Comuni di Abruzzo e Marche, salvando per loro la stagione sciistica. È

l'emendamento citato dal collega Ferrazzi del Partito Democratico è stato fatto saltare: meglio nulla ora, che una norma dannosa che avrebbe fatto fatto saltare il ciclo di quei rifiuti che tornano prodotti e che aveva allarmato non solo le imprese, ma anche le associazioni ambientaliste. Per gli enti locali, sono i milioni per gli investimenti ai Comuni e 250 milioni per la manutenzione di strade e scuole alle Province umiliate dal Governo Renzi nel 2014. Mi avvio alle conclusioni, ricordando che

come non citare le azioni fatte dal ministro dell'interno Salvini per garantire più sicurezza agli italiani e una gestione seria dell'immigrazione, che non solo ha bloccato gli sbarchi, ma ha fatto anche conseguire enormi risparmi nell'accoglienza, che ci consentono ora

per spuntare dalla Ue uno zero virgola di flessibilità ha svenduto il Paese, rischiando di trasformarlo in un campo profughi, firmando il piano operativo Triton, tenuto nascosto per tre anni al Parlamento, che - allora sì - è stato esautorato, non accettiamo lezioni. Non le accettiamo proprio.

provo tanta delusione e amarezza rispetto al metodo utilizzato per arrivare all'approvazione del più importante atto parlamentare e istituzionale che il Governo compie in quest'Aula. Mi riferisco naturalmente alla legge di bilancio che, detta così, sembra poca cosa, ma in realtà in essa è segnato il futuro di ciascun cittadino,

Avete urlato «onestà, onestà, onestà!» ma, una volta al Governo, avete voltato le spalle alla maggioranza degli italiani e alla democrazia del nostro Paese. Avete defenestrato proprio da quest'Aula quella democrazia che vi ha permesso di essere eletti portando in campagna elettorale le vostre promesse, naturalmente irrealizzabili, perché anche nel maxiemendamento che voterete in quest'Aula

e alcun emendamento presentato dagli altri Gruppi. Vi sfugge, però, un piccolo dettaglio molto importante; un dettaglio che fa emergere la vostra profonda contraddizione politica interna e che, soprattutto, vi delegittima a parlare a nome del popolo italiano. Voi non rappresentate la maggioranza dei cittadini italiani, né un Governo eletto dal popolo:

Questo vi impone un confronto politico sulla legge di bilancio, sia nel metodo che nel merito, con tutti noi che rappresentiamo quanti non vi hanno votato e che sono la maggioranza degli italiani. È vomitevole - permettetemi di dire - anche scorretto osservare come avete messo in discussione i princìpi della Costituzione che impongono un confronto nelle Aule preposte. Il vostro non è un cambiamento, non è un cambio di rotta con il passato, ma è semplicemente il risultato della vostra profonda contraddizione politica interna che, fino all'ultimo

chiaro, benissimo, ma raccontate la verità e dite a tutti che quella che chiamate *flat tax* riguarda fatturati fino a 65.000 euro. Avete annunciato la quota 100: bene, ottimo, ma dite la verità ai lavoratori, spiegando loro che potranno andare in pensione, ma avranno la decurtazione a vita di una parte della stessa pensione. Avete detto, affacciandovi al balcone di Palazzo Chigi, che avete abolito la povertà:

di più agli stranieri e a chi lavora in nero. Avete affermato di voler abolire la disoccupazione: bene, ma dite agli italiani che la legge di bilancio non prevede nulla per creare occupazione che il decreto dignità che avete approvato ha portato, secondo l'Istat, 36.000 nuovi disoccupati, e siamo soltanto all'inizio. State mandando a casa 5.500 lavoratori ex Lsu-Lpu in Calabria, oggi con il più alto tasso di disoccupazione. Avete annunciato il taglio delle pensioni d'oro: bene, ottimo l'annuncio, fantastico direi, ma dite agli italiani che le pensioni d'oro sono poche invece, avete penalizzato tutte le pensioni al di sopra dei 1.500 lordi con il blocco delle indicizzazioni. Avete colpito i lavoratori in pensione, non la casta, perché adesso siete diventati voi la casta. Avete festeggiato lo "spazzacorrotti": ottima la festa, ma raccontate ai cittadini che non avete atteso il parere del Consiglio superiore della magistratura arrivato in queste ore: un parere negativo, espresso a maggioranza schiacciante, con 17 voti a favore, compreso il voto di un vostro componente della maggioranza, tre contrari e astenuti; parere con il quale il CSM ha ribadito i rischi di incostituzionalità del vostro decreto. Per non parlare del manifesto dei 110 professori di diritto penale, il fior fiore dell'accademia italiana mai accaduta da quando esiste la nostra Repubblica - che si sono rivolti al presidente Mattarella come garante. Avete messo in allarme prima il mondo della sanità, mettendo in discussione la scienza con i vostri giudizi personali rispetto ai vaccini; adesso il mondo del diritto e delle libertà personali su cui si fonda il liberalismo democratico di tutto l'Occidente. Per finire, è in discussione il ruolo del Parlamento con la scelta di non discutere le proposte presentate da chi rappresenta - ribadisco - la maggioranza degli italiani, che sono quelli che non vi hanno votato. Avete annunciato che sarebbe stata la manovra del popolo e, invece, l'unica cosa che state cercando di manovrare è il popolo attraverso i vostri annunci irrealizzabili. Io ho piena fiducia, non in voi, ma nel popolo stesso perché sarà lo stesso popolo che vi ha votato che presto scenderà in piazza per mandarvi a casa. State facendo del male ai cittadini: oltre al gas e alla luce che sono aumentati dell'8 per cento, troveranno l'aumento dell'IVA sotto l'albero di natale, che arriverà per cento nel 2020. È una cosa improponibile; non è mai accaduto, nemmeno in Grecia. Per non parlare della TARI in bolletta che obbliga i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti assieme alla elettricità. Se questo non accade, la pena è il distacco della corrente elettrica. In che Paese vogliamo vivere? Vorrei spiegare ai cittadini che avremmo voluto parlare di *flat tax*, che nei nostri emendamenti si parlava di questo, dell'aumento delle pensioni, degli strumenti per creare lavoro al Sud, degli incentivi per le giovani madri, delle grandi opere, della TAV in Piemonte, della statale 106 delle tre Regioni, dei porti e degli aeroporti. Avete bocciato il Ponte sullo stretto, ma non vi siete preoccupati di mettere in sicurezza il porto che permette l'attraversamento dello dello Stretto di Messina, che è attraversato da 2 milioni di mezzi e che non è stato realizzato per questo traffico. Non avete accolto l'emendamento del porto e nemmeno quello dell'aeroporto di Reggio Calabria. Voi del MoVimento

nel vostro maxiemendamento. C'è soltanto l'elemosina: il reddito di cittadinanza. È una vergogna per il nostro Paese. I cittadini del Sud non si sentono di vivere con dignità in questo Paese. Potevate fare molto di più.

C'è poco da fare, le ricette che abbiamo avuto negli ultimi cinque anni - è inutile che ce lo nascondiamo - non hanno funzionato. Voglio evitare di ripetere cose già dette anche da me più volte, ma

FAZZOLARI *(FdI)*. È arrivato il Governo del cambiamento perché serviva un cambiamento. Peccato che il cambiamento non c'è stato perché la discussione surreale che abbiamo oggi è che la sinistra sta contestando una manovra che è in continuità con le sue manovre. State giocando in casa tra di voi. Questa manovra, infatti, ripete esattamente gli orrori e gli errori delle manovre degli ultimi cinque anni, non solo nei numeri. Il Governo del cambiamento era partito lancia in resta a dichiarare guerra all'Unione europea dicendo di

perché - un briciolo di conoscenze di macroeconomia potrebbero servire quando uno deve fare una manovra economica politiche espansive dal lato della domanda solo su spesa corrente non hanno mai funzionato nella storia delle economie occidentali; quindi, questa sarebbe stata la prima

saldi ancora peggiori di quelli previsti negli anni precedenti, quindi un *deficit* del 2 per cento e per di più interamente in spesa corrente. Ora, noi tifiamo sempre per l'Italia ma una brutta figura così mi chiedo perché l'abbiamo dovuta fare. Se si aveva l'intenzione di essere così poco il problema è che

per difenderla. Serviva una manovra sovranista. Che cos'è una manovra sovranista noi lo diciamo da sempre perché, per capirci, noi eravamo sovranisti prima ancora che questo termine diventasse di moda e chi scopre in tarda età di diventare sovranista, magari si confonde e non capisce esattamente di che cosa sta parlando. Una manovra sovranista è, ad esempio, quella fatta da Trump negli Stati Uniti: investimenti pubblici e riduzione delle tasse, anche pagata in *deficit* ma *deficit* interamente destinato a investimenti pubblici e riduzione delle tasse. I risultati si vedono e l'economia americana

sarà addirittura peggiore) vi sono 6 miliardi in più di tasse sulle imprese, e non sulle grandi perché almeno la metà di queste graveranno sulle PMI. Nessuna *flat tax* ovviamente, sempre dai numeri che avevamo finora, a fronte dei 18 miliardi in più di *deficit* per finanziare la spesa corrente, la spesa corrente, abbiamo solamente 3 miliardi in più per finanziare investimenti. Questo fa capire qual è l'orientamento di questa manovra. Oppure, una manovra sovranista è la manovra che stanno attuando i Paesi di Visegràd nella quale concentrano gran parte delle loro risorse al sostegno alle famiglie per un piano di natalità serio. Anche a questo proposito in questa manovra non c'è nulla. Una manovra sovranista avrebbe guardato all'unità territoriale della propria Nazione (mentre il divario Nord-Sud resta inaccettabile) e avrebbe concentrato le proprie risorse nel Sud, così come ad esempio ha fatto la Germania al momento della riunificazione, concentrando gran parte delle proprie risorse a riassorbire i territori dell'Est.

conclusione di una farsa era più che prevedibile. Beppe Grillo lo aveva annunciato anni fa, dicendo fieramente che grazie al MoVimento 5 Stelle in Italia non era cresciuta la destra. questo inganno per fortuna sta finendo. Con questa manovra abbiamo stabilito chi sono i sovranisti e chi può sfidare i tecnocrati di Bruxelles e non è certo questo Governo grillo-leghista ma solamente i sovranisti di Fratelli d'Italia.

siamo in Aula dall'altra notte con un dibattito assolutamente surreale: il Senato è impegnato a discutere di un testo che non c'è. Oggi, 21 dicembre, non abbiamo ancora un testo. Qualcuno di noi ha potuto leggere delle indiscrezioni sui giornali. Qualcuno ha potuto approfondire il maxiemendamento del Governo pervenuto in Commissione giustizia, ma chissà se poi sarà confermato nel testo del maxiemendamento del Governo. Abbiamo, quindi, solo anticipazioni dai giornali, quei giornali (e non stupitevi se io stamattina, come tutte le mattine, ho letto anche il *blog* di Francesco Storace), che voi volete tacitare, silenziare, chiudere e non finanziare più (ma su questo tornerò). Se il Senato fosse un teatro, se il Senato fosse un luogo di spettacolo, noi oggi saremmo spettatori di una grandissima opera del teatro italiano: «Questi fantasmi!», portati in Aula da Eduardo De Filippo. Sì, «Questi fantasmi!»", uno spettacolo reso famoso dal grande Eduardo, un testo nel quale, dietro l'apparizione di fantasmi, si nasconde la classica storia di un tradimento coniugale. Anche noi in Senato abbiamo da oggi dei fantasmi. Dei fantasmi nascosti dietro il ghigno del Sottosegretario presente in Aula dall'altra notte, che si trastulla con il suo *smartphone* per nascondere il fatto che si annoia e che ritiene inutile questo Parlamento, che ritiene inutile la nostra democrazia parlamentare, in scherno alla Costituzione e a tutto quanto in essa

gli attori europei di questo testo, che chissà se arriverà nel pomeriggio. Sono Juncker, Moscovici e Dombrovskis, i veri estensori della finanziaria che voteremo questa notte, con un voto di fiducia e quindi piegati, voi, pur se non la condividete, a dare ancora un respiro di ossigeno a questo strano Governo. Un testo scritto fuori dal Parlamento e negato alla conoscenza di ciascuno di noi. La Commissione bilancio non ha potuto votare nemmeno un emendamento. Ha esaminato un testo del tutto superato dal maxiemendamento del Governo, che chissà se arriverà. Siamo in Aula con lo spettacolo desolante di una legge di bilancio che arriva senza relatore, per la prima volta nella storia della Repubblica. E per la prima volta in assenza del presidente della Commissione bilancio.

se non si vergogna di essere la Commissione, si siede al banco delle Commissioni! Questa è la prova provata che, anche sulle Commissioni, voi avete messo una pietra tombale, sul luogo della democrazia e del confronto! Fatevi dare una lezione di Costituzione: state lì e metteteci la faccia. Metteteci la faccia!

Andiamo avanti sui contenuti, colleghi, quelli che non ci sono e ci dovrebbero essere. Purtroppo il presidente Pesco è andato ieri su tutti i giornali e vi è stata anche una sua dichiarazione; ha chiesto alla Presidente come poteva fare per andare avanti. Questo è il punto vero: come farà ad andare avanti, dentro la *pièce* di «questi fantasmi!», un matrimonio di comodo nel quale uno dei due coniugi è incatenato e non può mollare? Siete incatenati, perché avete il divieto di secondo mandato, perché sapete che siete in calo verticale, perché il coniuge più forte vi tiene inchiodati ai suoi interessi e, pian piano, vi mangia. Parliamo alla politica, di fatti, di quello che accadrà alle tasche degli italiani da domani notte.

è che a questi fantasmi ne mancano altri due; fantasmi qui dentro dal primo giorno, fantasmi da quando Conte è venuto a raccontare quelle quattro paroline che gli è stato concesso di dire sull'accordo con l'Europa. Abbiamo i due Vice *Premier* totalmente fantasmi, soprattutto nel loro ruolo. Uno crede di fare il Ministro dell'interno e si traveste: un giorno si traveste da poliziotto, un giorno da pompiere, un giorno da elicotterista*.

Abbiamo un altro fantasma, quello del Ministro del lavoro, che da oggi sarà il Ministro della disoccupazione e del precariato*. Che fatica che mi fate fare! Sarà il Ministro che ha tagliato la possibilità ai precari della pubblica amministrazione di essere assunti fino a novembre dell'anno prossimo. Questo vale anche per i precari dell'università e per tutti quei precari che aspettavano da tempo la loro stabilizzazione. Bisogna, allora, capire se, forse, forse, nell'essere fantasmi, avete scelto la sindrome del copiare. Infatti, proprio questa notte, il Ministro fantasma della disoccupazione ha scelto anche lui il travestimento (forse ha imparato da Salvini) e si è travestito da Berlusconi:

che questa falsa legge di bilancio, che nessuno ha potuto vedere, in realtà preoccupa la maggior parte degli italiani. Preoccupa chi deve provare a occuparsi del proprio futuro e del futuro dei propri figli.

partirà da "-23 per cento", che è quella clausola di salvaguardia sull'IVA che avete cercato di fermare oggi: aprite la porta all'austerità, a un'Italia sempre più precaria, sempre più sola, sempre più isolata continuate a farlo vergognandovi, perché di questo Governo oggi - poiché continuate con i fantasmi - non c'è nessuno.

Signor Presidente, il disegno di legge di bilancio per il 2019 rappresenta, con ogni

una situazione che sicuramente non ha precedenti. Siamo partiti, lo scorso mese, da un Governo che diceva «Me ne frego. Tiro dritto. Le letterine le lasciamo

Insomma, il Governo dei sovranisti è rimasto senza sovranità. Proviamo dunque a descrivere il testo, anzi, se mi permette signor Presidente, vorrei provare ad aggettivarlo: scialbo, inconcludente, annebbiato, strabico, inutile e, soprattutto, anche dannoso per il nostro Paese,

La manovra è stata talmente variabile, in questi giorni e in queste settimane, che nella maggior parte dei casi è sembrata è sembrata evanescente e soprattutto impercettibile. Dalla manovra di bilancio ci si aspetta anche una linea, una strada, una direzione, ma soprattutto una prospettiva, per invertire quello che è stato fino ad oggi un declino.

economica che in pratica scontenta tutti, dalle imprese alle famiglie, al mondo della scuola, a quello degli imprenditori, alle piccole medie e imprese, agli interventi per il Mezzogiorno. Non c'è un settore o un comparto della società civile o del mondo produttivo che esprima apprezzamenti per questa manovra economica, che ricordo è tutta finanziata con interventi di copertura a debito. Aggiungo che, anche per quanto riguarda l'ambiente, è stato fatto veramente poco. Tutto questo per non parlare delle ultime correzioni imposte, come dicevo prima, da Bruxelles, dopo il tira e molla

ovvero della revisione della clausola di salvaguardia. Ma come? Avete così criticato - e aggiungo che lo avete fatto giustamente - per tutta la scorsa legislatura l'introduzione della clausola di salvaguardia che rappresenta una misura sicuramente da non perseguire. Credo quindi che la legge di bilancio al nostro esame sia lo specchio vero e reale dell'inesperienza politica di questo Governo, impostata - non dimentichiamolo - su due capisaldi: da una parte il reddito di cittadinanza e dall'altra parte parte la quota 100, che non determineranno alcun impatto positivo sull'economia del Paese e anzi aggraveranno le tensioni

credo che questo braccio di ferro con l'Europa si sia risolto con un deprimente gioco dell'oca. A giudicare dalle reazioni soddisfatte e neanche troppo imbarazzate del Governo, è come se in questi ottantaquattro giorni non fosse successo nulla, come se durante il tempo trascorso tra la "notte del del balcone" ed oggi, tra la festa dello sforamento in *deficit*, con tanto di pugni alzati e dita in segno di vittoria e l'attuale ingloriosa retromarcia della manovra, l'economia italiana avesse aspettato alla finestra, tranquilla, senza subire un contraccolpo per i mesi

Altro che «abbiamo sconfitto la povertà»; il rischio vero è che con la vostra manovra purtroppo ci saranno ancora più poveri domani, ma soprattutto dopodomani, quando gli effetti della manovra si faranno sentire in tutta la loro negatività.

per me si deve fare tutto il *deficit* che è necessario. Il punto è che quando fai dei debiti, devi decidere anche che cosa ci vuoi fare con i soldi. Ecco, fare debito per fare spesa corrente non è mai una buona idea e non perché lo dica io.

siamo in una situazione di sovracapacità produttiva. Se mettiamo nelle tasche della gente 6.100 milioni di euro per fare spesa corrente, ciò non è sufficiente a costringere le aziende ad incrementare la produzione, fare nuovi capannoni ed investire su macchinari, perché hanno i magazzini pieni e siamo in sovracapacità. Quindi il moltiplicatore, che teoricamente sarebbe pari a uno, scende perché di questi soldi una parte definitivamente diverrà accumulo da parte del venditore di servizi o di prodotti; potrebbe quindi essere pari a 0,9 o 0,95. Ciò vuol dire che il rientro per lo Stato sarà inferiore.

Ho assistito per cinque anni alla genesi di ciò che viene chiamato reddito di cittadinanza che, più coerentemente, andrebbe chiamato «reddito minimo garantito condizionato». Inizialmente la cifra messa sul piatto era di 16.961 sarebbe andata per i centri per l'impiego e gli altri per finanziamento diretto, per una platea, stimata, ai tempi, di 9,5 milioni di persone.

(Rei); diventano così 3.950. Il paradosso è che si toglierà a qualche povero per dare a qualche altro povero perché le due platee di beneficiari non sono due insiemi perfettamente sovrapponibili; sono due insiemi con un'intersezione non vuota, ma con due bordini.

Statisticamente - per un attimo mi perdonerete il pollo di Trilussa - la divisione fa circa 90 euro a testa al mese. Questo vuol dire che qualcuno prenderà di più e qualcuno prenderà di meno, perché la somma è sempre quella. C'è chi prenderà 775 e c'è chi vedrà invece un assegno di 50. assegno di 50. Attenzione vorrei sollecitare sulle possibili criticità di un provvedimento di questo tipo: a fronte di questi, che possono andare da 1 a 779, viene chiesto un impegno mensile di trentadue ore per lavori socialmente utili. Diciamo che se ad una persona che prende 50 si chiedesse di lavorare per trentadue ore, vorrebbe dire che la sua retribuzione media oraria sarebbe pari a circa 1,51 euro all'ora. Mi sembra un *benchmark* salariale effettivamente molto risicato. Ma andiamo avanti:

dovrà gestire per lavori socialmente utili il 10 per cento della sua popolazione residente. Una città come Roma, che ha 2,8 milioni di abitanti, dovrà gestire 280.000 lavoratori socialmente utili. Come farà? Impossibile. Cosa gli farà fare? Gli farà fare quei lavori di bassa professionalità che vengono appaltati alle cooperative. A questo punto perché un Comune dovrebbe dare un appalto per il verde pubblico a una cooperativa, pagandola, quando c'è qualcuno che farebbe la stessa cosa pagato dallo Stato?

nel testo - che non so poi quale diventerà - erano originariamente scritte tre proposte di lavoro. Essendo buono e supponendo che siano mutuamente spendibili, sono 5,5 milioni di posti di lavoro, cioè si sta promettendo di crearne 5,5 milioni, ma siccome c'erano due vincoli (non più di 50 chilometri dal luogo di residenza al luogo di lavoro e non più di ottanta minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici), è chiaro che non possono essere 5,5 milioni: una persona che stesse a Santa Maria di Leuca non potrebbe accettare un lavoro a 51 chilometri di distanza. Entrando nel dettaglio (da matematico guardo il dettaglio, non mi interessa quando una funzione è olomorfa, ma mi interessa il punto di discontinuità), cosa intendiamo per mezzo di trasporto pubblico? Un mezzo di trasporto collettivo e non di proprietà: quindi un aereo o un treno ad alta velocità. Da Milano potrei allora essere costretto ad andare a Bologna: il treno ci mette meno di un'ora. Naturalmente, sono esclusi i tempi di percorrenza a piedi per il raggiungimento della postazione di presa del mezzo pubblico. Quindi, questi ottanta minuti non si sa quanti siano e non è comunque un criterio oggettivo. In ogni caso, non possiamo pensare di proporre a una persona un lavoro a 200 e oltre chilometri di distanza da casa propria, penso che saremo tutti d'accordo. Quindi, in realtà sono più di 5 milioni e mezzo di posti di lavoro. In teoria ci potrebbe anche stare, però - attenzione - i posti di lavoro in Italia li crea il privato. - dei posti di lavoro italiani sono creati dal privato. Quindi, lo Stato sta impegnando il privato a creare, lui, per il 75 per cento, almeno 5 milioni e mezzo di posti di lavoro: sono circa 4 milioni. Perché il privato crei posti di lavoro, sempre con i famosi moltiplicatori di prima, ci vogliono investimenti. Il privato deve essere incentivato a investire in filiera e piattaforma tecnologica per produrre nuovi posti di lavoro. Se gli investimenti non ci sono, il privato, sulla base di un mercato che non c'è, di una richiesta che non c'è e di un indirizzo politico che non c'è, cosa dovrebbe fare? Questo andrebbe bene in un'economia pianificata come la Cina, dove il Governo stabilisce cosa, come, dove ed entro quanto tempo e poi il resto si adegua. Questa è una cosa che qua non succede, quindi non è possibile fare un provvedimento di questo tipo senza l'altra gamba, cioè gli incentivi al settore produttivo. Sempre a proposito del reddito di cittadinanza, cosa dire ancora? L'Italia è una Nazione nella quale il lavoro nero prospera. Mi aspetto allora, come hanno fatto i prudenti finlandesi, una sperimentazione in piccolo per vedere quali sono le criticità e poi un'implementazione in grande, sempre che sia un provvedimento con le salvaguardie scalabili. Purtroppo, questo non è stato fatto quindi alla fine saremo noi le cavie e vedremo cosa andrà a succedere.

gli affidamenti diretti dei Comuni: erano 40.000 euro, adesso la soglia viene alzata a 200.000 euro, ma forse saranno 150.000 euro, che è pur sempre quasi quattro volte la soglia precedente. Premesso che io e altre persone qui abbiamo fatto battaglie colossali, dicendo che era il "marchettificio d'Italia" e che la soglia di affidamento a 40.000 euro andava abbassata, rifletterei anche su questo:

Questa era esattamente la cosa che per anni abbiamo combattuto, cioè impedire che il dirigente o l'assessore facessero un affidamento diretto a persone di loro fiducia: questo ora è dentro la manovra.

che devono spenderli le Regioni, con fondi propri. Beh, allora non hai messo 10 miliardi; hai ordinato a qualcun altro di spendere i soldi suoi su cose che decidi tu. Provvedimento giusto, ma almeno venditelo nel modo giusto; non vendertelo nel modo sbagliato.

chiudo - qui si è detto che l'Italia non è come una borsa o come un mercato finanziario. Però, vedete, non bisogna demonizzare né la borsa, né il mercato finanziario, perché è stata finora male interpretata. Il concetto è che nella borsa, che è stata tanto demonizzata, ci sono i fondi pensione e i fondi comuni, ci sono i soldi dei nostri

e dire che non fa niente se la borsa scende, perché sono tutti speculatori, significa darsi una mazzata. In questo contesto di regole dell'Unione europea, se tu vuoi andare allo scontro, non puoi prescindere dal fatto che loro vinceranno sempre. La via d'uscita, se a Monopoly non ti stai divertendo, non è provare a cambiare le regole, ma sedersi a un altro tavolo e giocare con altre regole. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membro del Governo, intervengo per esprimere tutti i dubbi, le perplessità e soprattutto le preoccupazioni, non solo del Gruppo di mia appartenenza (Forza Italia) tutta la maggioranza degli italiani, rispetto a questa manovra sciagurata proposta dal Governo giallo-verde. in questi ultimi giorni abbiamo assistito (in realtà l'Italia ha assistito) a uno spettacolo politico indecente, recitato da una maggioranza che non si è assolutamente rivelata all'altezza del compito che gli è stato affidato. Siamo stati prigionieri in quest'Aula e nelle aule delle Commissioni, in attesa di poter discutere di una manovra che non è mai arrivata né in Commissione, né ancora oggi in quest'Aula. Insomma, a regnare in questi giorni è stata l'assoluta confusione, fino ad arrivare a oggi, con una manovra ancora sconosciuta e che per di più arriverà blindata forse questo pomeriggio. Blindata da una fiducia che costringerà tutti noi a votare qualcosa che non conosciamo. Avete calpestato i diritti di questo Parlamento, quei diritti che fino a qualche mese fa, colleghi dei 5 Stelle, facevate finta di difendere e che oggi avete calpestato con una *nonchalance* imbarazzante. Siamo in definitiva al sovvertimento delle regole della democrazia. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una manovra su cui non sarà possibile intervenire, una manovra scritta e riscritta sotto dettatura dell'Europa. Una magra, magrissima figura per chi, dal primo giorno, si era tolto la maglietta e aveva fatto finta di mostrare dei muscoli inesistenti e che oggi, invece, è costretto a subire le bacchettate dell'Europa. Siamo qui riuniti ad apprendere questo ennesimo fallimento del Governo. Io, così come tutti i colleghi della minoranza, ma penso anche della maggioranza, in questi mesi ho lavorato per contribuire a scrivere degli emendamenti che potessero migliorare questa legge finanziaria. Avremmo voluto discutere ed entrare nel merito di tutti gli emendamenti; magari poi, come diceva ieri il collega Vitale, vederli respinti, ma almeno poterne discutere. Invece no, con l'imposizione della fiducia, voi membri del Governo avete impedito ad ogni

fatte dagli esponenti 5 Stelle si traducessero in provvedimenti concreti, in misure che potessero realmente migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, soprattutto del Sud.

Ho aspettato che questo emendamento, come lei aveva detto, fosse presentato nel decreto-legge Genova e non ne ho visto l'ombra; ho aspettato che fosse presentato nel decreto fiscale e non ne ho visto l'ombra; ho aspettato che fosse presentato nella manovra finanziaria Grazie

Del resto, per il Sud, per la Calabria in questa manovra non c'è assolutamente nulla. Penso ancor di più alla ministra Lezzi, che non più di quattro o cinque giorni fa è venuta a fare visita, la solita passerella, in Calabria, per dire che ci sarebbero stati dei finanziamenti, degli aiuti per le zone colpite. Ministro Lezzi, anche lei ha preso in giro per l'ennesima volta i cittadini calabresi. Se avesse voluto rispettare quello che ha detto non più di cinque giorni fa, aveva l'occasione di poterlo fare oggi; invece, anche in questo caso, si ha un fallimento. I grillini quindi hanno fatto solo parole, solo fumo, e preso per il naso non solo i calabresi, ma tutti gli italiani. Avevo presentato, come ogni collega (ma ci tengo a parlare di ciò avevo presentato io), qualche emendamento che potesse aiutare il Sud. Avevo pensato, per esempio, ad una proposta che prevedeva una riduzione delle tasse per tutte le aziende che nasceranno nel 2019 nel Sud Italia, perché questo serve al Meridione, non il reddito di cittadinanza, non l'umiliazione di una mancetta per stare a casa. Avevo preparato un altro emendamento che poteva concedere alle Province in dissesto di ripianare i debiti, non in cinque anni ma in dieci, però non sarà possibile discuterne. Avevo previsto, insieme alla collega Gallone, un emendamento che potesse dare agevolazioni fiscali a tutte le imprese che volevano investire nei centri dell'entroterra italiano, alle prese con il crescente fenomeno dello spopolamento.

La invito a concludere, senatore sono i nostri figli, le future generazioni che si ritroveranno a pagare i debiti accumulati da questo Esecutivo. Questa è la realtà delle cose. Questa è la situazione disastrosa in cui ci troviamo, ma a voi membri del Governo questo dramma non sembra interessare.

giorno e notte e non inutilmente, perché il maxiemendamento che arriverà è scritto non sotto dettatura, ma sulla base di quanto è stato discusso e del confronto che ha coinvolto anche l'opposizione. Da due giorni sentiamo interventi che sono più simili ai commenti di quei tifosi frustrati che, non potendo sperare nella vittoria della propria squadra, sperano nella sconfitta della squadra rivale, soprattutto quando gioca in Europa.

E di sangue i cittadini italiani ne hanno versato parecchio, sul piano economico. Due cose vere però l'ha dette persino lui. Quanto

in questo Governo ci sono gli unici partiti che non hanno responsabilità per i disastri degli ultimi sette anni, che si sono riversati sulla pelle dei cittadini e sono i quali - e lo vorrei ricordare ai colleghi Ferro e Verducci - è vero che a noi sono stati 2 miliardi di garanzie perché, come Paese, siamo cattivi pagatori, ma il problema è che cattivi pagatori di promesse sono stati loro e le garanzie dobbiamo metterle noi.

che si chiama Achille Marigo, ha scritto al sindaco di Rocca Pietore qualche settimana fa, dopo i disastri. Il bambino ha scritto: sono Achille Marigo, nove anni, abito a Mira, mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto, vorrei rivedere montagne con i boschi, perché da grande mi piacerebbe entrare

e non per contare, poi, i danni e i morti. Concludo dicendo che le regole, anche quelle europee, hanno senso se vengono applicate in maniera intelligente, flessibile e rispettosa della volontà democratica: alla fine, l'ha dovuto riconoscere in conferenza stampa perfino Moscovici. Sono regole di buonsenso, che il 4 marzo, con il voto degli italiani, abbiamo portato nel Parlamento italiano e che a maggio contiamo di portare in quello europeo, con altrettanto

Signor Presidente, negli scorsi mesi abbiamo sentito più volte il Governo, e in particolare il ministro Salvini, intervenire sui temi della sicurezza, facendoli diventare una priorità, spesso legata al tema

rimandiamo a casa gli immigrati irregolari clandestini (più di 500.000); aiutiamoli a casa loro. Sono una persona che ama controllare le cifre e i numeri,

un momento in cui la nostra società, e in particolare quella italiana, vive una delle sfide più grandi dal punto di vista demografico, ossia la denatalità, mentre la sponda Sud del Mediterraneo, soprattutto l'Africa, conosce

fino allo 0,27 nel 2016, quindi con i Governi Renzi, e, da ultimo, allo 0,30 con il Governo Gentiloni Silveri. La Nota di aggiornamento al DEF

2030, su cui ci siamo impegnati come Governi europei all'interno delle Nazioni Unite. Ci siamo invece risvegliati con una doccia fredda, perché, nel documento della legge di bilancio, dei 5,8 miliardi promessi nella Nota di aggiornamento ne abbiamo solo 5, ben 800 milioni in meno: per la prima volta, dopo un *trend* positivo, ritorniamo sotto lo 0,3 e quell'«aiutiamoli a casa loro» diventa solo lo *slogan* da

miliardi è gestito direttamente dal Ministero dell'interno: non sono soldi che vengono utilizzati per la cooperazione allo sviluppo, ma sono soldi che vengono utilizzati per i richiedenti asilo. ed era iniziato un dibattito in questo senso - se vogliamo veramente rimandare gli immigrati irregolari nei loro Paesi, quei soldi devono essere utilizzati meglio. La mia preoccupazione è che quei soldi, invece, vengano messi, non sui rimpatri volontari assistiti, come avevamo iniziato a fare con i nostri Governi, ma sui rimpatri forzati,

di riammissione, che faticano a funzionare. Il più importante è l'accordo con la Tunisia e noi abbiamo trovato un modo molto bello per farlo funzionare: la prima dichiarazione del ministro Salvini è

Le cose invece funzionerebbero, se utilizzassimo quei soldi per rimpatri volontari assistiti legati a progetti di cooperazione. Certo, serve collaborare con le organizzazioni non governative e serve destinare una parte di quel miliardo alla creazione di occasioni di autoimprenditorialità non bastasse, con questa manovra assistiamo per la prima volta al taglio dei finanziamenti al sistema delle Nazioni Unite. Ancora una volta, se si vogliono fare i rimpatri

che già sarebbe una giustificazione fondamentale necessaria e sufficiente - ma ha a che fare anche con la sicurezza del Paese: 1,250

Le persone che scappano da lì e i Paesi di origine non hanno alcun interesse a fare gli accordi bilaterali di riammissione, perché chi è qua manda le rimesse e, se accendessimo un attimo la testa e pensassimo al nostro passato, durante il secondo dopoguerra mondiale

Gli *slogan* di cui dicevo all'inizio servono magari per prendere qualche voto in più, per vincere qualche ballottaggio, ma non per vincere le sfide decisive, quelle della cooperazione allo sviluppo, del finanziamento alle organizzazioni internazionali, del finanziamento ai rimpatri volontari assistiti che potremmo cominciare a chiamare in maniera diversa e della collaborazione con le organizzazioni non governative,

potremo governare nell'immediato, ma non risolveremo i problemi dell'Italia e, soprattutto, non daremo una speranza di futuro a chi sta in quel continente, che continuerà a guardare ai Paesi europei come il punto di riferimento e il luogo in cui arrivare. Cambiamo atteggiamento e proviamo ad andare oltre l'immediato, per tentare di dare una visione strategica, non solo alla nostra politica estera, ma alla politica economica e della cooperazione allo sviluppo del nostro Paese.

e direbbe: dove sono finiti tutti i professori e gli opinionisti che hanno calcato tutti i *talk show* in questi anni raccontando di un'Europa matrigna, le loro tesi economiche, come avrebbero fatto loro una volta arrivati al Governo per far rispettare la sovranità italiana? Questa occasione l'avete avuta; ce l'avete e non mi pare, visto l'andamento del dibattito tra l'opinione pubblica, che la continuiate a portare avanti. Si sono tutti defilati, sono tutti *desaparecidos*. Parlando con alcuni di loro ho potuto constatare il rammarico del fallimento delle loro tesi nel momento in cui dovevano attuarle. Poi sapere cosa si chiederebbe questo fantastico marziano? Ne è valsa la pena di sei mesi di insulti e di scontro frontale con l'Unione europea?

per tutti questi anni e oggi alcuni colleghi della maggioranza si congratulano tra di loro perché da 300 è arrivato a 250. Come cambiano le cose; cambiano sempre, purtroppo, in peggio. Ora

ha comportato il risultato strategico del Governo del cambiamento. Qualcuno della maggioranza ci ha spiegato che è un negoziato: quando si negozia parte e controparte piccola notazione: quando si negozia, l'imprenditore pensa al suo patrimonio e ai suoi soldi, voi avete negoziato mettendo le mani nelle tasche tasche e avete preso i soldi dei risparmiatori italiani. Tutta questa roba l'avete fatta con questa modalità, non con i soldi vostri, ma con i risparmi e le imprese italiane.

Dico poi una cosa che veramente mi ha lasciato di sasso: avete ridotto del 50 per cento l'Ires a tutte le strutture del terzo settore, anche a quelle di culto che non hanno fine di lucro. Noi - lo voglio dire con estrema chiarezza, amici della maggioranza - siamo da quella parte, siamo a sostegno di quei volontari che con passione, sacrificio e umanità si dedicano al prossimo. Quei servizi integrano il Servizio sanitario nazionale e non vanno in competizione e voi avete ridotto per cento. Per non parlare del reddito di cittadinanza: non voglio utilizzare le parole del sottosegretario Giorgetti, ma permettetemi di dire che finalmente qualcuno comincia a dire la verità. Lui l'ha definito: non serve a nulla e crea lavoro nero. Non l'ha detto un esponente dell'opposizione, l'ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se non siete d'accordo, allora ribellatevi; se non siete d'accordo con la trattativa che questo Governo ha condotto con l'Unione europea andate avanti, siate coraggiosi, portate avanti le vostre tesi, se ci credete, altrimenti tutto ciò sembra una pantomima. Nel momento in cui dovevate sbattere i pugni siete tornati indietro con la coda fra le gambe. Signor Presidente, non è un regalo di Natale allora questo, anzi, chiedo scusa, è un grande pacco di Natale. Anche in questo caso vorrei citare un film che forse ricorderete, un grande film: «Regalo di Natale» di Pupi Avati,

che in questi anni ha fomentato l'alternativa (e forse qualcuno si è anche pentito), perché ritenevate gli altri non credibili, non adeguati e talvolta corrotti.

troppo monopolio. Attenzione, cari amici, perché le bugie si misurano con la realtà è presto la realtà diventerà verità e i consensi si ridurranno, come si sono ridotti per chi vi ha preceduto. Presidente, mi permetta di chiudere parafrasando una citazione

tra la guerra all'Unione europea e il disonore. Avete scelto il disonore e avete chiesto scusa all'Unione europea. *(Applausi

io forse vi stupirò per come voglio iniziare questo mio intervento, che segue i brillanti interventi, tecnici e specifici, dei miei colleghi che già nelle ore precedenti, nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, hanno avuto modo di evidenziare l'incongruenza economico-finanziaria di questa manovra della quale voi vi assumete la totale paternità. paternità. Intervengo in questo momento innanzitutto per elogiare la coerenza di una delle forze politiche che guida questo Governo. Intervengo per elogiare, amici a 5 Stelle, e lo faccio senza ipocrisia alcuna, la vostra coerenza. Ricordo delle piacevolissime conversazioni con il vostro mentore, con il comico Grillo, con il quale ho condiviso anni in ristoranti e in un ameno albergo romano e con il quale spesso mi intrattenevo negli anni passati a dialogare e a discutere. Devo dire, però, che mai avrei pensato che quelle affermazioni, che il simpatico comico genovese portava al tavolo, fossero poi, in realtà, un pensiero politico che si sarebbe tradotto in atti parlamentari. Egli ha tentato tante volte, con la sua simpatia, di convincermi che il reddito di cittadinanza sarebbe stato il futuro di questo Paese. Mi diceva sempre che la dinamica industriale avrebbe portato al fatto che la maggioranza del popolo non avesse lavoro, che tutti dovessimo prepararci a stare a casa e che, quindi, lo Stato doveva darci da vivere. Questo è quello che mi raccontava e io lo ascoltavo, sempre pensando e ricordando qual era il suo vero ruolo e qual era la sua vera attività, cioè quella del comico. E devo dire che mi divertivo anche. A distanza di qualche anno, però, il Movimento che da lui è nato e che a lui si ispira ha concretizzato queste parole: la decrescita felice. la decrescita felice. Guardo gli amici ed alleati della Lega, con i quali nelle piazze abbiamo parlato e continuiamo insieme a parlare, agli imprenditori, di crescita. Ebbene, la decrescita felice non è altro che la base filosofica e concettuale, cari colleghi, che ha improntato e impronta questa manovra economica. Ecco perché, senza ironia e con assoluta sincerità, io elogio fermamente la coerenza del MoVimento 5.

c'è una manovra che è arrivata qui in Senato, sulla quale non abbiamo avuto modo di lavorare in Commissione, dove non abbiamo avuto modo di esprimere un solo voto, manovra che è stata poi completamente stravolta e che, magari, può essere ancora parzialmente modificata con il superemendamento della fiducia, che conosceremo, auspico, nel pomeriggio. Quindi, non è tanto sulla manovra in sé, quanto su un percorso che io voglio fare la mia analisi. Un percorso che nasce, come ho detto, prima concettualmente, a livello personale, da Grillo, ma che nasce, a livello parlamentare, già questa primavera, quando si è cominciato a parlare del DEF, quando siamo arrivati al decreto dignità, quando dal decreto dignità siamo arrivati alla Nota di aggiornamento del DEF, quando dalla Nota di aggiornamento del DEF siamo arrivati al decreto fiscale e, quindi, alla legge di bilancio quale essa sarà. Ebbene, in tutti questi documenti e normative cosa abbiamo letto? Cosa possiamo leggere da questa documentazione? Intanto, una assoluta mancanza di sensibilità alle istanze che ci sono pervenute e che ci pervengono quotidianamente dalle categorie. Siete riusciti, cari amici della maggioranza, a far arrabbiare

per arrivare ai miei colleghi dottori commercialisti: in sostanza, quel mondo che produce e al quale, cari colleghi, non frega un bel niente - passatemi il termine - del reddito di cittadinanza, ma che vorrebbe meno imposte, vorrebbe un fisco migliore e più chiaro, vorrebbe una giustizia diversa. Quelle categorie che lavorano e che volevano che quei miliardi, che voi destinate al reddito di cittadinanza, fossero investiti per rendere i nostri tribunali più più agevoli e più utilizzabili e non tribunali che aspettano dieci anni per emettere una sentenza, non commissioni tributarie che, di fatto, sono l'inaffidabilità assoluta per chi se ne intende di diritto tributario. tributario. O nel cuneo fiscale, che appesantisce i nostri lavoratori rispetto ai lavoratori del resto del Paese. Queste sono le risposte che la classe produttiva si attendeva da noi. Ecco perché, dalla grande finanza, dagli industriali, arrivando ai piccoli imprenditori, agli artigiani e ai tassisti sono tutti arrabbiati e noi siamo arrabbiati con loro. Questa è l'analisi del vostro comportamento politico di questi mesi. Questa è un'analisi impietosa che, purtroppo, trascinerà il Paese nella recessione. questa manovra, cari amici, cari colleghi, signor Presidente, signori del Governo, e lo sapete voi prima di me, state facendo il conto del tempo che vi separa dalle elezioni europee.

a petto in fuori e che invece vi ha visti protagonisti, in modo miserevole, di una cedevolezza assoluta. Io avevo detto in quest'Aula al presidente Conte, di andare a Bruxelles a testa alta, magari di modificare qualcosa in quella manovra, ma di non farsela dettare da Bruxelles. Qual è stato il risultato, cari colleghi? Che mentre Bruxelles dettava elegantemente la manovra ai colleghi del Partito Democratico, a voi l'ha imposta arrogantemente, ridicolizzando questo Paese.

questo. Signor Presidente, mi conceda ancora un minuto. Voglio anche ricordare che c'erano tante possibilità di cambiare la manovra, perché noi non siamo coloro che criticano. L'opposizione patriottica della destra italiana (perché noi siamo la destra coerente, la destra che è da sempre italiana e per gli italiani) vi aveva fatto delle proposte nel merito. Ci era stato

assistenzialismo, per far arrabbiare gli imprenditori e i commercianti, ma non c'è stato tempo per rispondere alle proposte di crescita che Fratelli d'Italia, coerentemente con la propria vocazione, aveva fatto. Concludo, Presidente, ricordando che avevate a disposizione gli 80 euro, quegli 80 euro che voi per primi, insieme a noi, avete irriso e condannato perché avevano creato una discriminazione sociale tra lavoratori autonomi e dipendenti; avevate a disposizione quel denaro per per fare anche crescita e non lo avete utilizzato, neppure quello. Ebbene, la condanna che voglio rivolgere alla politica che ha ispirato la vostra manovra finanziaria è assoluta e totale.

esame certifica un grande *bluff*, il primo grande fallimento del contratto di Governo, che si poneva ambizioni nel cambiare il Paese, l'Europa, la società, l'economia. Nella realtà, quando uscirete da quest'Aula, anche dopo il voto di fiducia, capirete che questa manovra compromette il futuro e colpisce al cuore le speranze e le aspettative degli italiani. Tagliate le pensioni, bloccando l'indicizzazione delle stesse; aumentate le tasse per le imprese: sono tagli alla spesa, quelli che voi chiamate rimodulazioni, e sono nuovo gettito fiscale. Ma, inevitabilmente, queste due misure contrarranno i consumi e soprattutto gli investimenti. Spingete le famiglie italiane verso forme di nuova povertà e il tutto avviene, colleghi, all'interno di comunità più individuali, dunque più fragili e più deboli. Promuovete ogni giorno, culturalmente, con i vostri messaggi, il «me ne frego», anziché il «me ne occupo» tra i cittadini. Il «ci pensiamo noi», anziché il «facciamo insieme con l'azione di Governo». Separate il pubblico dal privato, la società dal mercato, il capitale dal lavoro, individuando ovunque nemici e avversari. Colleghi senatori, abbiamo idee e programmi profondamente alternativi e differenti sul piano valoriale e culturale. Abbiamo presentato, attraverso i nostri emendamenti, una manovra alternativa, dimostrando che si poteva, con il buon senso e la razionalità, coniugare una buona gestione dei conti pubblici con un più forte sostegno alla crescita e allo sviluppo. Infatti, senza spingere la crescita non ci sono le condizioni strutturali per ridurre le disuguaglianze, attraverso un nuovo investimento sui servizi, sul *welfare*, dunque sulle persone e sui diritti delle stesse. Avremmo orientato oltre 2 miliardi di euro verso il reddito di inclusione e avremmo modificato la legge Fornero in maniera selettiva, partendo dalle donne e dai lavori usuranti:

avremmo ridotto il costo del lavoro, per aumentare i salari, garantendo alle imprese sgravi fiscali nell'assunzione dei lavoratori veri, delle persone. Questa sarebbe stata la misura fondamentale per attrarre crescita e sviluppo. La nostra contromanovra, però, non è stata affrontata e discussa.

che vi ha imposto una retromarcia, che tuttavia, colleghi, per la prima volta compiete senza il popolo. È infatti una retromarcia senza il popolo e onerosa per il popolo, perché è costata oltre 1,5 miliardi di euro solo per la gestione del debito, per la mania sovranista di aprire un conflitto per ragioni di consenso, senza alcuno sbocco e senza alcuna visione per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Avete isolato l'Italia in Europa e avete tardivamente corretto questa impostazione. Avete portato voi, non noi, l'Italia a rischio di un'infrazione sul debito, grazie all'instabilità, all'arroganza e soprattutto al sovranismo, che vi impone un conflitto per mantenere il consenso. Avete scelto i sussidi, con una promessa per tutti: ai disoccupati avete promesso un reddito, agli evasori un condono, ai lavoratori l'abolizione della legge Fornero, ai cittadini italiani avete promesso di rimandare a casa propria i clandestini. È però tutto il contrario di quello che state generando. State generando infatti nuova solitudine e nuova indifferenza, state riducendo la propensione agli investimenti, state spingendo gli investimenti L'Italia, anche se muscolarmente appare solida e certa nelle mani del Governo, è in realtà più debole e più insicura e ci troveremo più clandestini e meno sicurezza. Gruppo PD)*. Agite sugli individui con la propaganda, dimenticando che esiste una comunità di persone che chiede, nella dignità, lavoro e crescita, ma soprattutto futuro e speranza per i nostri figli. Avete annunciato e festeggiato l'abolizione della povertà, senza una legge e senza un decreto. Un annuncio fine a se stesso, dimenticando che la prima misura universale per contrastare la povertà è il reddito di inclusione, che noi abbiamo realizzato e che voi trovate già nel bilancio dello Stato. In questa manovra

quelle parrocchie, quegli oratori e quei contenitori sociali che da sempre sono al lavoro per aiutare le persone e che, nei fatti, sottraggono la povertà alla solitudine e all'indifferenza. Questo

perché se vogliamo contrastare la povertà, non lo possiamo fare per decreto, ma con un'alleanza nel territorio, tra l'associazionismo e il volontariato. Deve tornare protagonista il «me ne occupo», oltre che le risorse necessarie per garantire un servizio e un reddito. Ci siamo chiesti più volte se tutto questo sia il frutto di una superficialità o di un'improvvisazione. Penso il contrario, ovvero che sia una strategia politica e il volto del sovranismo, che si è radicato anche nel sentimento degli italiani. Avete bisogno del rancore, della rabbia, vi servono i conflitti e avete bisogno di sterilizzare e di congelare il rancore e la rabbia per gestire il consenso. Non volete trasformare questa rabbia e questo rancore in speranza, perché cadrebbero il populismo e il sovranismo. Così, cari colleghi, uccidete però il futuro dell'Italia e compromettete la crescita e la propensione agli investimenti, unica leva fondamentale per dare ai giovani un futuro migliore. A pagare purtroppo il conto salato delle vostre iniziative sono gli italiani; sono già stati i risparmiatori e gli imprenditori, che oggi faticano più di prima ad attrarre nuovi investimenti ed avere un accesso al credito utile per generare nuovi investimenti. Siamo invece di fronte a curve, sopratutto sull'accesso al credito, negative e restrittive per le imprese. Anche la scelta operata nella legge di bilancio di concentrare tutto in un rapporto esclusivo tra il Governo e la Commissione europea, addirittura negando al Parlamento gli atti fondamentali che stanno alla base di quella relazione, è un colpo gravissimo alla democrazia. È un colpo favorevole a dare l'idea che state lavorando sottotraccia, in solitudine, senza il coraggio di dire agli italiani cosa si anche all'interno dell'accordo che avete compiuto e delle misure di verifica, alle quali l'Italia verrà sottoposta ulteriormente dall'Europa. È soprattutto un rapporto diretto tra il Governo e il popolo, saltando il Parlamento.

deboli di fronte ai conflitti, a perdere è l'intero Paese. Fate in modo di recuperare la credibilità delle Istituzioni e della democrazia perché essa serve a garantire un futuro al Paese. Anziché qualificare la democrazia con la partecipazione, mettete il bavaglio all'editoria. Cancellate, per cortesia, questi tagli; sono vergognosi e limitano la libertà di informazione e la possibilità nei territori di conoscere, di leggere, di sapere di interessarsi e di occuparsi della comunità nella quale vivono. Non sono costi, ma investimenti per la cultura, per la conoscenza e per il futuro di una comunità.

Una manovra che scarica 23 miliardi nelle clausole di salvaguardia compromette il futuro. L'Italia non è nelle condizioni di reggere oggi la manovra del 2020-2021. Colleghi, attenzione perché fare queste operazioni significa rendere impraticabili lo sviluppo e la crescita economica e portare l'Italia ad essere il Paese in Europa con l'IVA più alta. In questo modo si contraggono i consumi

cercate di ascoltare e monitorare attentamente l'attuazione della manovra che sarà difficile, complessa e impatterà in un ciclo economico che per il momento non ci mette nelle condizioni di avere un Governo pronto per affrontare una nuova sfida. Cambiate la manovra

Signor Presidente, ieri un assistente parlamentare mi ha accolto dicendomi che avevo un meraviglioso sorriso e sembravo felice. Gli ho risposto che non ero felice, ma raggiante perché stavo assistendo ad una cosa che se avessi potuto crederla vera, avrebbe rappresentato una svolta nella vita politica del

perché sarebbe forse la prima volta dal 1494 (quando Ludovico il Moro, come sappiamo, chiamò Carlo VIII per risolvere un piccolo problema di politica interna) che si depone in questo Paese la prassi di chiamare una potenza estera in proprio soccorso per risolvere problemi interni. Di questa prassi - va detto - il PD è stato negli ultimi anni, lo dico oggettivamente, autorevole interprete: «ce lo chiede l'Europa» o «ce lo chiedono i mercati» è stato il grido di battaglia che abbiamo sentito risuonare tante volte, mentre i nostri autorevoli e competenti interlocutori politici si scagliavano all'assalto dello Stato sociale, della scuola, della piccola e media impresa e delle istituzioni che costituivano e costituiscono la spina dorsale del Paese, sempre con il sostegno di un'Unione estera che per ovvi motivi non poteva più essere quella sovietica, ma - pur cambiando aggettivo - la subalternità non era cambiata. anche l'attitudine critica verso l'Europa che vediamo oggi non è un'assoluta novità. «Se restiamo fermi, prigionieri di regolamenti e burocrazia, l'Europa è finita»: chi ha detto queste parole? Un sovranista? No, un *leader* dell'attuale opposizione, che ha trovato un rifugio nel ramo del Parlamento che un tempo voleva abolire e che oggi ci chiede di rispettare. Anche noi vogliamo rispettare questo ramo del Parlamento. *(Applausi dai è che vorrei che fossimo oggettivi e sereni nel riconoscere che la compressione del tempo del dibattito non è dipesa da noi, ma dipende da un insieme di regole esogene che finora sono andate bene alle opposizioni, perché sono servite per scaricare

mette sempre più in luce la deriva antidemocratica che il progetto ha preso. Naturalmente gli elettori assistono a questi strepiti e si chiedono: chi ci ha portato in queste condizioni? *(Applausi dai Gruppi

in realtà ha fatto sul serio una cosa che prima di noi i Governi precedenti avevano fatto solo a chiacchiere, quando avevano la vera possibilità di agire. Ha negoziato con l'Europa, ha negoziato sul serio e senza compromettere l'interesse del Paese, come qui è stato più volte ripetuto. Ha anche fatto un'opera di misericordia, che è visitare gli ammalati, perché l'Unione europea è profondamente malata e bastano pochi esempi a metterlo in evidenza. È chiaro che si sarebbe potuto ottenere di più. Certo, in ogni negoziato serio si può ottenere di più. Ci si può sempre comportare in modo migliore e noi siamo sempre disposti ad ascoltare i consigli di chi non può più dare cattivo esempio, come già ricordato in altra sede. Intanto quello che è accaduto ha messo in evidenza l'assurdità delle regole europee, in particolare il loro carattere prociclico. Ci è stato detto che le nostre previsioni di crescita erano sbagliate e abbiamo dovuto fare previsioni più realistiche. La verità è diversa e quello è uno snodo tecnico.

il cosiddetto *output gap*, senza il quale l'Europa non ci avrebbe magnanimamente concesso di disporre di più risorse per rianimare il Paese. Purtroppo il problema è che se ti chiedono di diminuire la crescita, le risorse sono in quota di quella crescita e quindi alla fine l'Europa ti costringe a fare uno sforzo con risorse inferiori rispetto alla necessità. Questi sono i miracoli di un meccanismo opaco e assurdo, nonché scientificamente infondato. Sarebbe stato meglio, allora, tenersi la regola del 3 per cento sul saldo nominale, quella regola che Prodi definitiva stupida, ma che aveva due vantaggi: quella di essere trasparente e verificabile, due cose molto importanti in democrazia, perché qui stiamo parlando di previsioni, di ipotesi e di molteplici stime e su questo siamo ipotecando il futuro del nostro Paese. I fatti, invece, dimostrano che le regole dei trattati l'Europa può permettersele. La famosa regola del 3 per cento del rapporto fra saldo di bilancio nominale e PIL nominale l'Italia se la può permettere. Sapete chi l'ha violata di più fra i grandi Paesi europei? Naturalmente in testa abbiamo Grecia e Portogallo, le cui economie sono state martoriate dalla crisi. Ma poi, con 13 violazioni, segue la Francia; e 11 di queste violazioni sono consecutive. Caro Presidente, le do una notizia fresca: il commissario Oettinger ha chiesto che venga aperta una procedura di infrazione contro

Questo, forse, è l'unico argomento che avrei accettato dall'opposizione: dato che i conflitti stavano per emergere ed era così evidente che stavano emergendo, questo avrebbe consigliato un atteggiamento più prudente, aspettando che gli altri si combattessero fra loro, in questa meravigliosa famiglia europea, senza dare loro pretesti per attribuire a noi delle criticità che non dipendono da noi. È stato molto interessante ieri sentire qualcuno citare BlackRock, che sconsiglia agli investitori di comprare i BTP. Ora, il salto da Marx a BlackRock è abbastanza ardito, ma è soprattutto molto significativo. Pochi giorni fa, infatti, «Il Sole 24 Ore» ci riferiva che questa importante società di consulenza è stata la capofila fra le società che hanno gestito, a botte di decine di milioni, gli *stress test* sulle banche europee.

viene attribuito il compito di garantire il merito di credito dei nostri istituti. Questo è il risultato di riforme fatte in fretta; riforme ambiziose, certo, ma che sono state fatte senza il necessario consenso politico e senza le risorse e gli strumenti necessari. Che una moneta unica implicasse una vigilanza unica doveva essere chiaro fin dall'inizio; non si doveva poi correre ai ripari con dei consulenti, che hanno fatto quello che hanno potuto, per carità. Vi rendete perfettamente conto di cosa significa affidare a chi specula sui titoli bancari il compito di valutarne il merito. Questa cosa è talmente assurda, che vi dico un secondo conflitto franco-tedesco: Schäuble, che non è esattamente un nostro amico, ha chiesto conto dell'accaduto alla signora Nouy, per sapere se ci fosse già evidenza di fughe di notizie e di conflitti di interessi. Questa è la BCE, l'istituzione che pochi giorni fa un autorevole economista, Donato Masciandaro, definiva "il faro nelle nebbie", un faro talmente efficiente che non riesce neanche a seguire la rotta che lui stesso indica, perché noi l'inflazione al 2 per cento, che ci avrebbe aiutato ad alleviare il carico del nostro peso, non l'abbiamo vista. Abbiamo la deflazione e ancora si dispera

c'è un interessante comma, che serve a rimediare a uno dei tanti disastri fatti a colpi di decreto e sfuggiti alla vigilanza unica. Ed è quello che si sarebbe verificato, se noi non fossimo intervenuti, con i gruppi bancari cooperativi, voluti dall'attuale

Questo è il risultato delle riforme fatte in fretta e questo è il risultato della vigilanza che vigila solo quello che interessa a lei di vigilare. D'accordo? Queste sono le nostre asimmetrie. E voglio dire che non è facile ovviare a questo e ad altri disastri sparsi nelle pieghe del nostro ordinamento, a questi treni lanciati in corsa, sempre per dimostrare di arrivare prima degli altri, per ovviare a un complesso altri, per ovviare a un complesso di inferiorità che i nostri cittadini non sentono più e del quale voi vi siete fatti in qualche modo interpreti, mettendo il Paese in condizioni di seria e oggettiva difficoltà. A questo aggiungerei un'altra misura contenuta nella manovra: permettere alle piccole banche di adottare principi contabili più confacenti al loro modello di *business*, come succede in tutta Europa, come succede in particolare in Germania. Piace la Germania? E allora facciamo come in Germania. Come ha fatto la Germania? Ha violato la regola del 3 per cento sette volte (noi otto) e le sue banche hanno i principi contabili nazionali. Beh, da questa manovra in poi, anche le nostre piccole banche potranno avere la stessa facoltà.

cambierà la musica anche lassù e la prossima manovra verrà negoziata con interlocutori più attenti agli interessi dei singoli Paesi. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tratterò del conflitto franco-tedesco, della pace di Aquisgrana o di non so che altro, perché non sono professore universitario

Il collega Bagnai dice che c'è stato un *deficit* di subalternità, ma voi siete la quintessenza della subalternità all'Europa con quello che è successo in questi giorni. Io ne ho viste tante di manovre, di maxiemendamenti, di fiducie e credo anche il presidente Calderoli come me, quindi mi meraviglio poco, ma stavolta mi sono meravigliato anche io. Ci avete tenuto in ostaggio in Senato, non si è votato nemmeno un emendamento e diciamo al Presidente della Repubblica di vigilare sulla violazione dell'articolo 72 della Costituzione. FI-BP)*. È molto grave, infatti, che la Commissione bilancio e il Senato non possano discutere la manovra, ma Moscovici e Juncker ve la possono dettare fino nei dettagli. Altro che *deficit* di subalternità:

indecorosa, incostituzionale e gravissima. Non si è votato un emendamento in Commissione bilancio. L'incolpevole Presidente della Commissione bilancio, privo di esperienza, ha chiesto: che devo fare, Presidente? Una persona che ha una responsabilità applichi le regole e la Costituzione; non venga qui a chiedere cosa deve fare.

perché il presidente del Parlamento europeo Tajani, quando Juncker ha straparlato nell'Aula di Strasburgo, lo ha messo a posto, non ha fatto lo scribacchino come Conte e come altri. se volete lezioni di orgoglio italiano, ve le possiamo offrire gratis*.* Avete truffato sulle cifre relative al *deficit* e sul reddito di cittadinanza. Delle due l'una: la cifra è tagliata a 6 miliardi, perché un miliardo va ai centri per l'impiego. Se i poveri che ne hanno diritto, ai quali noi guardiamo con grande rispetto, sono 6 milioni, la divisione dei 6 miliardi per queste persone dà

Avete fatto danni ai disabili e voglio dire che in Parlamento non c'è la caccia al parlamentare, c'è la vergogna per voi che avete costretto dei parlamentari ad abbandonarvi perché avete bocciato le proposte per i disabili. *(Applausi

Questo avete fatto: il blocco delle pensioni da 1.000 euro netti. Il Paese sappia che questo Governo blocca le pensioni dei poveri e fa poi la propaganda su altre. La *flat tax* è scomparsa. Noi, con il programma del centrodestra, con coerenza sosteniamo *flat tax* per tutti e non la piccola truffa che avete fatto per pochissimi.

Gruppo FI-BP).* Questa è la verità. E il vostro precedente decreto dignità fa scomparire, ogni ora del giorno o della notte, 26 posti di lavoro. È il decreto povertà, altro che il balcone! Questa manovra ha colpito perfino gli oratori. La manovra sull'Ires colpisce associazioni, imprese e oratori. Ieri anche la Conferenza episcopale italiana vi ha dovuto bacchettare, perché avete mortificato anche chi non fa speculazione commerciale, ma gestisce delle attività per raccogliere persone che si radunano. Avete ridotto le agevolazioni per le imprese, cancellato una serie di benefici fiscali e fuori manovra

Avete massacrato la sicurezza e le Forze armate, perché volete ridurre i militari a tappa buche per la Raggi. Non consentiremo questa vergogna! *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Chiediamo scusa, a nome vostro, ai militari italiani che lavorano per la nostra sicurezza in patria e all'estero, non devono andare a bitumare le strade che devono essere gestite dai Comuni. Se la Raggi non è capace, si dimetta e non invochi le Forze armate!

L'elenco dei massacrati è enorme. Alcuni se ne sono accorti, altri se ne accorgeranno. Nella conferenza stampa che la presidente Bernini ha tenuto poco fa è stato detto che state tartassando tutti. Il collega Giro mi suggerisce un *cadeau* a Conte: il film «I tartassati», con Totò e

missive. Per una settimana i colleghi della Commissione bilancio non sapevano di cosa discutere. Volevamo risposte sul trasporto pubblico e privato e sui balneari. Vi chiediamo di essere concreti. Forza Italia chiede che per alcune categorie - balneari e ambulanti - ci siano risposte immediate. Alzate la testa contro l'Europa, come noi vi chiediamo e come quest'Assemblea ha deliberato, su proposta di Forza Italia, il 27 giugno scorso, chiedendo la tutela di quelle categorie! Cari colleghi, non ci siamo: l'avvocato del popolo si è rivelato uno stenografo di Juncker, ma noi siamo Forza Italia e vi voteremo contro in nome del popolo italiano.

del Governo, è surreale ascoltare le opposizioni parlare del mancato dibattito sulla legge di bilancio. Mi ricordo

E ora sento parlare di dignità del Parlamento: non siete credibili e, così facendo, lo sarete ancor meno. Vorrei fare un po' di storia, perché in due giorni ho sentito parlare tanto di queste clausole di salvaguardia sull'IVA, come se le avessimo messe noi. Senatore Marcucci, vedo che mi aiuta a tenere ordine nel Gruppo.

Poi, nel 2013, il Governo Letta aumenta l'IVA dal 21 al 22 e sposta le altre clausole. Funziona così: anno per anno si vanno a sterilizzare le clausole di salvaguardia, che è quanto stiamo facendo noi; ma noi non lo possiamo fare, perché... GIRO non spetta a lei fare il correttore delle bozze: se la senatrice commette errori, sicuramente in buona fede, finisce lì. Senatore Airola, è il momento di andare a fare un giretto alla *buvette*: vada

e gli italiani a un altro bilancio, su un'altra strada. Peccato che questa strada, nonostante il passaggio dal Governo Monti ai Governi Letta, Renzi e Gentiloni

che andavano contro i cittadini ma a favore delle *lobby*, abbiamo deciso di fare un'altra manovra stiamo cercando di salvare il Paese, un Paese che ha più di 5 milioni di poveri, che ha una popolazione anziana che, com'è stato ricordato, non si può curare o non accende il riscaldamento.

degli incentivi per le *start-up*, perché crediamo che quello sia il modo giusto per far crescere il Paese.

tutti i cittadini avevano bisogno e continuano ad aver bisogno del reddito di cittadinanza, il vecchio Governo targato PD introdusse il Rei, ossia la brutta copia del reddito di cittadinanza, diciamolo. *(Applausi Avete una narrazione tutta vostra, riuscendo a vedere le cose e a raccontarvele come volete.

avete raccontato un Paese e una storia tutta vostra, partendo già dalla riforma della Costituzione. Ricordo i titoli dei giornali in cui si prevedevano catastrofi, se avesse vinto il no: ha vinto il no

che siamo dovuti andare in Commissione europea a riconquistare la fiducia. Tutto quello che avete fatto voi fino ad oggi è stato distruggere il Paese, non solo moralmente, ma anche nella fiducia che gli altri Paesi avevano

Senatore Verducci,

In questa Aula sentivo parlare di strategia, noi l'abbiamo fatta una strategia. Avete portato il Paese sempre in emergenza e i crolli dei ponti non sono colpa nostra, ma ci stiamo pensando noi.

che loro ci offendano. Cara senatrice Bottici, lei che è stata la principale attrice della confusione e della violenza in questa Aula, non ci violenza in questa Aula, non ci venga a dare lezioni. Le macchiette non siamo noi, siete voi una macchia per il Paese intero. Si vergogni di offendere i colleghi.

quello che lei ha riferito. Ci sono delle frasi che verranno sicuramente sanzionate; altrimenti ci troveremmo di fronte a un caso di calunnia. Verificheremo chi dei due ha realizzato questi comportamenti.

Signor Presidente, senatrici e senatori, vorrei ringraziare sinceramente i senatori e le senatrici della Commissione bilancio che con pazienza hanno seguito i lavori in questa fase convulsa. Avrete modo di notare che numerosissime istanze dei Gruppi verranno accolte proprio perché

il reddito di cittadinanza e la quota 100, di cui si è dibattuto ampiamente, così come non entreremo nel merito degli ultimi emendamenti perché, come spesso accade quando si valuta una manovra, si guarda l'ultimo miglio e ci si dimentica di quello che sta dietro. Ci concentreremo, dunque, nel dare risposta ai tanti interventi di ieri sera e di oggi, su due argomenti in particolare, cioè il tema relativo agli investimenti e il tema sociale. Ora, la considerazione di fondo che muove questa manovra è la come mai, nonostante una congiuntura astrale particolarmente favorevole - il petrolio ai minimi, i tassi di interesse ai minimi, il QE, l'espansione monetaria di Draghi

regole contabili, burocrazia, la scelta di fare sempre cose nuove e dimenticarsi della manutenzione straordinaria e il contenzioso con gli enti locali. regole contabili, per gli enti territoriali e per i comuni era impossibile spendere liberamente l'avanzo di amministrazione. Con una circolare della ragioneria abbiamo tolto questo vincolo per cui dall'anno prossimo, anzi già da quest'anno, tutti i comuni d'Italia possono spendere liberamente l'avanzo di amministrazione. Solo questo comporta circa un miliardo di investimenti aggiuntivi in più. burocrazia, il codice degli appalti, fatto con le migliori intenzioni del mondo, ha però bloccato la spesa di investimento in maniera importante,

quei piccoli investimenti diffusi in tutto il Paese che consentono una ripartenza più veloce del PIL, investimenti che hanno un doppio beneficio: innanzitutto la veloce spendibilità perché sono di piccolo importo e poi, soprattutto, le asfaltature non si importano per cui, grazie a questi piccoli investimenti, riempito di *gilet* arancioni, che sono un po' meglio di quelli gialli, e sono i *gilet* delle nostre aziende che ritorneranno a fare un po' di lavoro.

sostegno diffusa su tutto il territorio e per tutti i Comuni di media e piccola dimensione, siamo convinti si riesca a far ripartire un po' il PIL, soprattutto nel settore costruzioni. manutenzione, anche in questo caso la scelta di chiamare attorno a un tavolo le maggiori aziende pubbliche consente di far ripartire molto più velocemente la spesa. Faccio un esempio. La sola ANAS ha a bilancio circa un miliardo di euro per la manutenzione straordinaria. Banalmente, raddoppiare da un miliardo a due miliardi, nello stesso *budget* esistente nell'ambito della società, la manutenzione straordinaria consente di far ripartire moltissimi cantieri, anche qui in tutto il Paese, in tempi molto rapidi. Vi è poi il tema del contenzioso con gli enti territoriali. Di quei 150 miliardi già esistenti, cui si aggiungono i circa cento appostati con il disegno di legge di bilancio, di investimenti legati all'attività sul territorio, circa ottanta erano bloccati per un contenzioso con le Regioni. Semplicemente chiamando le Regioni attorno a un tavolo noi abbiamo chiuso un accordo in Conferenza Stato-Regioni e sbloccato oltre ottanta miliardi, che erano appunto bloccati per un contenzioso. È questione di mettersi attorno a un tavolo e discutere con gli enti territoriali, cosa che negli ultimi anni era diventata un po' difficoltosa. Si era preferito il muro contro muro e un certo rapporto di centralizzazione, e non di dialogo, con gli enti territoriali.

una buona parte del sociale. Ci si dimentica, nel guardare la manovra, che sono stati appostati oltre 500 milioni di euro in più sul sociale, oltre mezzo miliardo in più. 123 milioni aggiuntivi sul fondo della non autosufficienza. *(Applausi dai sul fondo famiglie e disabili, che non esisteva. Sono cento milioni per il fondo disabilità e famiglia, che non esisteva, messi a decorrere, cioè non per un anno ma per sempre. 120 milioni aggiuntivi sul fondo delle politiche sociali: aggiuntivi.

Si tratta di interventi molto importanti nel sociale, di cui si sente parlare poco. Il mezzo miliardo aggiuntivo, però, va anche considerato in relazione al reddito di cittadinanza. Mi spiego.

Questa spesa si troverà, quindi, libera per nuovi interventi, poiché la maggior parte della platea insiste ancora sul reddito di cittadinanza, favorendo così una diffusione maggiore di questo *welfare* di comunità, necessario soprattutto in ambito dell'integrazione socio-sanitaria, che sappiamo essere uno dei temi più importanti del futuro della nostra Nazione. Parliamo, quindi, appunto di sanità. Nonostante tutte le difficoltà del caso, il fondo sanitario aumenta di 4,5 miliardi nel triennio ma soprattutto, e anche questa misura è stata poco sottolineata, sono stati stanziati quattro miliardi di euro aggiuntivi di di investimenti in edilizia sanitaria, cosa di cui c'è una enorme necessità nel nostro Paese. Quindi, questi sono anche investimenti particolarmente mirati su un settore che ha bisogno di un'assistenza particolare.

Sviluppo e detassazione delle aziende: sappiamo che le due cose vanno di pari passo. Per avere sviluppo abbiamo bisogno di investimenti e anche di meno tasse; questo è ovvio e, soprattutto, è opportuno e normale in un momento in cui il mondo sta andando da quella parte. Se si va verso una detassazione in tanti Paesi, anche noi dobbiamo muoverci in quella direzione. Non è semplice in questo contesto, ciononostante sono stati fatti degli interventi importanti. Il primo, il più noto, è quello che riguarda le partite IVA più piccole. È un tema assolutamente rilevante, perché aver esteso il regime dei minimi a 65.000 euro (c'è poi la parte da 65.000 a 100.000 euro al 20

la terza valenza di questa misura, che spesso viene sottovalutata, è la potenzialità di emersione del sommerso che oggettivamente ha. Diciamoci le cose come stanno. Noi abbiamo aree del Paese in cui vi è un tasso di disoccupazione giovanile con percentuali abnormi; ove non ci fosse l'attività cosiddetta informale avremmo la rivoluzione: non c'è la rivoluzione perché c'è attività informale, sostanzialmente il lavoro nero. Il regime dei minimi è anche uno strumento molto efficace per far emergere finalmente, in tante realtà, lavoro che c'è e che semplicemente non viene denunciato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo è un punto fondamentale, che dobbiamo sottolineare, di questa misura. Oltre a questo, sono stati fatti altri interventi, ma non mi voglio dilungare troppo. L'ultimo è la riduzione dei premi INAIL, che era attesa da anni;

Per non parlare del raddoppio della detassazione dell'IMU sui capannoni: anche questa è una misura molto sentita, soprattutto dagli imprenditori medio-piccoli.

Per i Comuni, oltre alle questioni classiche, abbiamo introdotto un fondo sul modello spagnolo, per dare una forte spinta agli investimenti e, a fianco di questo, la semplificazione del codice degli appalti: è tanta roba, aggiunta allo sblocco totale della spesa dell'avanzo di amministrazione. Per le Province vi è il riconoscimento della dignità di un ente che si voleva cancellato, che il popolo sovrano ha deciso rimanesse e che purtroppo era totalmente definanziato, le strutture peggio messe nel nostro Paese sono le due strutture in capo alle Province: gli istituti scolastici superiori e le strade provinciali.

il Paese. Quei 250 milioni di euro a decorrere sono un segnale molto importante in questa direzione, a cui si aggiungono altri fondi di investimento, che vedremo poi nel dettaglio. Infine, per le Regioni abbiamo raggiunto un'intesa importante su diversi temi. Abbiamo parlato prima del tema sanitario; allegato a questo c'è il tema dei contratti. Ci si dimentica - ma penso sia importante rilevarlo in questa sede - che l'accordo che abbiamo concluso con le Regioni ha evitato il taglio di 1,4 miliardi di euro sui fondi delle politiche sociali. Non autosufficienza, fondo delle politiche sociali, libri di testo, fondo per i disabili: questi fondi sarebbero stati cancellati se non si fosse trovata una soluzione. Ebbene, non solo abbiamo trovato una soluzione, eliminando 1,4 miliardi di euro di tagli, ma abbiamo

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Ai sensi dell'articolo 129, commi 2 e 3 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Dopo la votazione degli

si procederà alla discussione dell'articolo 1 del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Sarà quindi posta in votazione la Nota di variazioni e si procederà infine al voto del disegno di legge di bilancio nel suo complesso. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge e nella Nota di variazioni. Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 2 a 19). In relazione agli emendamenti riferiti alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio, la Presidenza dichiara inammissibili, analogamente a quanto già stabilito durante l'esame in 5a Commissione, gli emendamenti 9.0.1, 10.1 e 12.1.

il Governo vuole scrivere da solo questa legge di bilancio; e allora la scriva e ci presenti l'emendamento sui cui porre la fiducia. Visto che non è stato disturbato da voti della Commissione i voti che abbiamo espresso adesso davvero non dovrebbero disturbare la serenità di coloro che stanno scrivendo (parte sotto dettatura di Bruxelles e parte con altri criteri) la nuova legge di bilancio, sarebbe logico che il Governo si presentasse qui con il maxiemendamento oppure che si andasse avanti a votare gli emendamenti, come dovrebbe essere e come si è sempre fatto nel passato.

Non vorrei che ci trovassimo di nuovo in un percorso. Quindi chiederei di avere una conferma.

essere dubbi sul fatto che alle 16 sarà presentato il maxiemendamento, anche perché il rappresentante del Governo poc'anzi ha rappresentato all'Assemblea una situazione che era evidente

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato i tempi della discussione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo della prima sezione della legge di bilancio.

La discussione sulla fiducia, per la quale sono state ripartite circa quattro ore in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà luogo a partire dalle ore 16, dopo la pronuncia da parte del Presidente sull'ammissibilità dell'emendamento sulla base del parere della 5a Commissione permanente.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato altresì, all'unanimità, il calendario dei lavori dal 9 al 17 gennaio. *(Commenti dal Gruppo PD).* L'Assemblea riprenderà i propri lavori mercoledì 9 gennaio, Gruppo PD)*, con la discussione della Ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale e di altre ratifiche di accordi internazionali concluse dal Gruppo PD)*, i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e il disegno di legge sulla videosorveglianza, ove concluso dalla Commissione.

Cosa vi siete venduti, colleghi, che non siete capaci, non avete il coraggio di dire ai vostri elettori? Vi siete venduti i pensionati italiani? *(Applausi

tempo, di convincere i pensionati che hanno più di 1.300 euro netti al mese che sono dei pensionati d'oro? *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. È per questo che ci state facendo aspettare? State cercando di convincere gli italiani che un reddito di cittadinanza di 83 euro al mese è tale e

di fronte a questo fallimento, di fronte a questa vergognosa manifestazione di incapacità e di dilettantismo da parte di un Governo che deve decidere le sorti di tutti noi, noi non possiamo tacere. Noi possiamo solo cercare di fare la nostra parte. Ci abbiamo provato fino adesso, ma non abbiamo mai avuto possibilità di parlare. Avete umiliato e imbavagliato il Parlamento, avete umiliato e imbavagliato il popolo FI-BP e PD)*. Gli italiani che vi stanno guardando, i pensionati che saranno impoveriti dal vostro Governo, tutti gli italiani a cui aumenterete le tasse e abbasserete

poi alle 11, poi alle 12, poi alle 14 un maxiemendamento che, per la vostra incapacità, proprio non riuscite a partorire. Evidentemente avete da fare i conti con l'Europa; questo Governo del questo Governo del vero duro, che si è presentato in Europa per spezzarle le reni ed è ritornato a casa con la coda tra le gambe, dopo aver tentato di fare puro *deficit* italiano, garantito dai suoi amici sovranisti, adesso evidentemente ha qualche problema con l'Europa, oltre che con la Ragioneria generale dello Stato. non fate pagare tutto questo agli italiani. Non fatelo pagare più di quanto abbiate fatto finora. È un cinepanettone che agli italiani costerà ben più del prezzo del biglietto di quello che si sta proiettando adesso nelle sale italiane. PD)*. Ben più di 8 euro costerà agli italiani questo cinepanettone vergognoso! Chiediamo dunque che l'Assemblea si riconvochi domenica, per discutere seriamente, quando il maxiemendamento sarà presentato, prima in Commissione e poi in Davanti agli italiani, colleghi del Governo e della maggioranza, abbiate il coraggio di farvi vedere. Siete diventati quelli che in Commissione bilancio hanno negato lo *streaming* per non farvi vedere all'opera dagli italiani

fate concludere la senatrice Bernini. impegnatevi tutti perché questo maxiemendamento esca. Metteteci in condizione di lavorarci sopra nell'interesse del Paese e domenica, con serietà, votiamolo tutti insieme: voi voterete a favore e vi assumerete le vostre responsabilità; noi voteremo contro, ma facciamo una cosa seria agli occhi del Paese. Avete già fatto cose abbastanza ridicole. Adesso, colleghi, vi prego: basta!

le difficoltà del Governo, che ci sono state anche in relazione all'interlocuzione con l'Europa, mi corre l'obbligo di invitare la maggioranza e il Governo ad avere un percorso legislativo

*(PD)*. Signor Presidente, mi ha fatto piacere la sua presa di posizione chiara. Ero rimasto perplesso prima, quando ci diceva che non capiva su cosa si stesse protestando. Mi sembra evidente su cosa si stia protestando:

I tre Sottosegretari presenti sono sicuramente adeguati e autorevoli, ma credo che il momento sia grave per la democrazia e per la Repubblica. Però loro non avevano tempo da dedicare al Senato. Sa perché, signor Presidente? Ce lo spiega il presidente Conte, Conte, con un'agenzia che è uscita in questi minuti, alla quale forse lei dovrebbe replicare. Il Presidente del Consiglio purtroppo non controlla il Parlamento: questo ha comunicato, giustificando il fatto che non abbiamo ancora votato. Non ha avuto il coraggio di dire che la vergogna del Governo è quella di non essere stato ancora in grado di portarci qua una manovra. *(A**pplausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. Non abbiamo nessuna informazione sulla manovra che saremo obbligati a votare. È una vergogna e il presidente Conte a questo aggiunge la beffa, signor Presidente, che lei non può più permettere, perché il diritto di ospitalità c'è tra galantuomini

Signor Presidente, se questo dovesse avvenire, se domani il presidente Conte dovesse essere in sala Koch a vantarsi della manovra

È ora di farla finita di umiliare le istituzioni. È ora di farla finita. Siamo entrati, signor Presidente, nella riunione dei Capigruppo con la proposta del ministro Fraccaro - nel frattempo anche lui è andato a fare *shopping* perché, come tutti sappiamo, siamo vicini al Natale e non poteva essere presente con noi in ci ha garantito che la manovra non sarebbe stata presentata alle 16, come previsto oggi, ma alle 8 domattina. Abbiamo posto qualche dubbio e allora ci ha garantito che sarebbe stata presentata domani mattina alle 9,30. A fronte poi di una nostra perplessità, percepita dalle nostre parole e dalle nostre espressioni, ha detto che forse l'avrebbe presentata alle 12. Poi, quando abbiamo chiesto di proporre il calendario, sono apparse le 14. Però vogliono votare domani. si sono presi due mesi per umiliare il Parlamento e il Paese; si sono presi due mesi per andare a Bruxelles a farsi dettare la manovra.

si devono capire e chi scrive deve sapere quello che scrive. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Evidentemente il nostro Governo, che si è fatto dettare la manovra, non capisce oppure non sa scrivere, tanto che sono giorni che siamo qua ad aspettare. signor Presidente, ci hanno preso in giro e ci continuano a prendere in giro, ma hanno la pretesa che si rispettino i loro tempi, hanno la pretesa di fare in modo che il Parlamento e il Senato votino una manovra senza poterla capire, approfondire e leggere.

lo faremo quando ne discuteremo. Una manovra sbagliata, pericolosa e drammatica per il nostro Paese. Non entro dentro la manovra; entro, come spesso mi capita in questa Assemblea, a difesa di questa istituzione e del Parlamento, contro il MoVimento 5 Stelle e la Lega

l'atteggiamento del Governo, la violenza che ci hanno fatto anche poco fa, sono pesanti. Signor Presidente, chiediamo a lei e a tutta la Presidenza, chiediamo agli autorevoli colleghi di dire basta a questo modo di procedere. Ve lo chiediamo per favore! Abbiamo bisogno del vostro aiuto per difendere le istituzioni. Non è possibile accettare questo calendario. Noi abbiamo proposto dall'inizio una cosa semplice. Qualsiasi fosse il momento nel quale veniva presentata la manovra, ci fosse dato il tempo di leggerla e approfondirla. Le sembra troppo, signor Presidente? Le sembra troppo che il Senato abbia il tempo di votare con cognizione di causa, con scienza e coscienza? Non è troppo, è il minimo. E oggi non ci viene garantito neanche il minimo. È un attacco vergognoso alla democrazia di forze politiche che lavorano contro l'Italia e contro la democrazia. Noi voteremo no al calendario.

abbiamo assistito, come lei sa, ad una riunione dei Capigruppo ancora una volta abbastanza speciale.

Per questo avete preso

cosa ancora? L'umiliazione non ha più limite. Noi siamo costretti a vederne una dietro l'altra. Guardate, non venite a dire che ne abbiamo già viste. Di fiducie ne abbiamo viste tante; di ritardi di maxiemendamenti ne abbiamo visti tanti, ma siamo visti tanti, ma siamo ostaggio da giorni e giorni. La Commissione bilancio è stata ostaggio per più di due settimane con un Presidente che non sapeva cosa accadeva e nessuno che era in grado di mantenere una cosa che aveva promesso. Avevano detto i tempi, ma niente: nessun tempo è stato rispettato. Avevamo chiesto, anche

come tempo per presentare il maxiemendamento. Con la discussione, come si vede, siamo arrivati alle ore 14. Io penso, come ho sostenuto alla Conferenza dei Capigruppo, che ognuno di noi si assume le proprie responsabilità. La maggioranza e il Governo si devono assumere le loro responsabilità: hanno detto adesso le ore 14, ma ho paura che sarà un'altra volta una presa in giro. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo avere tutto il tempo; la Commissione deve vedere bene tutto, se mai sarà presentato questo maxiemendamento. Pertanto, per quanto ci riguarda, non esiste niente: si va a oltranza, perché dobbiamo avere la possibilità di poter vedere quello che c'è in questa manovra. Aggiungo un'altra cosa. Abbiamo fatto un'altra domanda al Governo. chiesto di spiegarci quali sarebbero queste ragioni tecniche che stanno ritardando la presentazione del maxiemendamento. Sappiamo tutti che non sono motivazioni tecniche. Forse c'è un problema di copertura di qualche misura? Ancora state litigando

che ho l'onore di presiedere. È stata una pazienza infinita e un senso di responsabilità infinito. Voi state rischiando di portare il Paese all'esercizio provvisorio *(Applausi

trasporto: siamo in una situazione kafkiana. Anzi, vorrei scomodare una citazione: «Aspettando Godot». Tutti la conoscono, è un'opera teatrale di Beckett che si associa al dramma dell'assurdo e al teatro dell'assurdo e che

noi siamo qui di rinvio in rinvio. Il maxiemendamento oggi non c'è, non è arrivato per le ore 16 stabilite; il calendario è saltato. Nella Conferenza dei Capigruppo, dove abbiamo fatto e disfatto il calendario, cercando di trovare tutti la soluzione migliore per il Paese (non per le nostre vacanze), alla fine dobbiamo dire ci è stato replicato e spiegato, in modo laconico, che questioni tecniche rinviavano l'arrivo del maxiemendamento. Ci sono sempre questioni tecniche, lo sappiamo bene. Ci sono sempre questioni tecniche, ma ci sono anche - dobbiamo dirlo, dovete dirlo, dovete ammetterlo - questioni politiche. Voglio anche dire che, di rinvio in rinvio, rinvio, qua si sfiora una situazione di esercizio provvisorio, perché si rischia di non approvare la manovra, finché non arriva il maxiemendamento. Perché la questione è politica? Perché evidentemente bisogna armonizzare gli *slogan* e le cose urlate nelle piazze con le coperture che non ci sono; ma soprattutto perché c'è da armonizzare il ritocchino europeo. Questo è il punto e il nodo politico. I tecnici devono oggi trovare una quadra rispetto al ritocchino di Bruxelles, perché non ci nascondiamo che di questa manovra ne sa più Bruxelles che questo Parlamento italiano;

una quadra. La manovra del popolo non decolla, ma in compenso il popolo vi guarda e rimane incredulo rispetto a quello che si sta verificando. Increduli siamo anche noi, che per senso di responsabilità

da lì nasce il ritardo. Noi per senso di responsabilità siamo stati in quella Commissione e siamo presenti in quest'Aula, perché per noi viene prima di tutto il Paese. Noi al Paese una manovra gliela vogliamo dare, una manovra giusta. Questi rinvii e questa pantomima alla quale ci state facendo abituare - ma non ci vogliamo abituare e non ci abitueremo - sono la metafora plastica, plastica, estetica e politica delle contraddizioni di un Governo, di quel corpaccione che dicevo prima, che si ostina a stare insieme barcollando tra un sovranismo che non riesce a esprimere e un globalismo dall'altra parte che rimane soffocato. Siete una somma di contraddizioni e queste contraddizioni nella manovra finanziaria esplodono tutte, perché i nodi vengono al pettine. E allora, vedete, se non ce la fate e se non avete il tempo,

siamo qui, ma vorremmo vedere linearità, coerenza e capacità di incidere e di produrre. Producetela questa manovra, cercate i tempi e i modi. Noi a questo calendario siamo contrari, perché è evidente che c'è una dilazione di tempi che non siete in grado di governare (sottolineo governare) e non siete in grado di controllare. E non è colpa dei tecnici, ma delle vostre contraddizioni politiche.

la Presidente sia testimone del fatto che nella Conferenza dei Capigruppo il clima è sempre costruttivo e sereno da parte delle forze di maggioranza e ancor di più da parte delle forze di opposizione. Poi in questi giorni ho sentito molte cose, molte accuse, ho sentito parlare di *unicum* nella storia della Repubblica; allora qualche qualche ora fa mi sono preso un po' di tempo, perché ero desideroso di valutare se veramente stavamo facendo cose mai accadute; mi sono preso delle ore perché pensavo di dover tornare almeno agli anni Sessanta,

Dopo di che sono arretrato di qualche anno e ho visto quello che è successo nel 2014, quello che è successo nel 2014, quando, dopo ore di rinvii, in quest'Aula è stata posta la fiducia alle ore 19, è stata votata la manovra alle ore 5 del mattino ed è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo alle ore 7 per calendarizzare l'Italicum e questo accadeva quattro anni fa,

sono perfettamente consapevole che c'è una situazione complessa legata al fatto che appena mercoledì l'Europa ha sciolto le riserve su un'eventuale proceduta d'infrazione, che siamo riusciti ad evitare tenendo insieme i conti, quindi le esigenze di bilancio con le esigenze sociali di questo Paese,

dovuto, e a nostro giudizio da esso giustificato, al negoziato europeo, che si è concluso proprio pochi giorni fa. Vi è quindi una ragione di questo tipo,

rispetto al copia e incolla del fax di Bruxelles a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. ci vuole tempo e la Ragioneria non era abituata. Questo è il motivo!

per annunciare il comportamento del nostro Gruppo rispetto al voto sulle proposte alternative che sono state avanzate rispetto al calendario votato a maggioranza dalla Conferenza

Riteniamo vergognoso, offensivo e sconcio nei confronti degli italiani continuare a rimandare il momento in cui questo Senato, rappresentante di tutti gli italiani, potrà leggere una manovra che si annuncia di lacrime e sangue, contro i pensionati, i giovani

Presidente, è un tema importante. Noi le chiediamo attenzione su questa vicenda, in quanto ne va della dignità del Senato. Chi umilia e offende il Senato della Repubblica non può qui avere ospitalità e noi ce ne faremo carico. *(Applausi

di drammatiche, certo non così dilettantistiche, ma ce ne sono state molte anche in passato. Quello che mi ha meravigliato - e dopo le dico come voteremo - è l'orgoglio con cui il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha rivendicato

una situazione identica al passato - lo dico con rispetto - è la tomba di quel cambiamento che avevate promesso, sempre che

non si è capito perché, dopo essersi riuniti - probabilmente per accorciare i tempi della lite, immagino io - hanno deciso di farci fare domani un *tour de force* senza darci il tempo di

questo programma. Lo facciamo senza iattanza, colleghi; non stiamo né urlando né insultando. Stiamo semplicemente dicendo che per un'opposizione patriottica, quale quella che abbiamo cercato di fare ora, è dura continuare a essere patriottici di fronte a un Governo che di patriottico non ha veramente nulla.

Faccio presente che rappresentanti del Governo, in sede di Commissione bilancio, avevano detto che l'emendamento era pronto si stava aspettando solo la lettera della Commissione europea. Così ci avevate detto. Lo aveva detto anche un Sottosegretario in Conferenza dei Capigruppo. Per una Per una questione di rispetto di questa Assemblea, di cui lei, Presidente, è garante, è giusto

Perché dobbiamo leggere sulla stampa cosa c'è o meno all'interno della manovra? Questa istituzione non sa nulla di vero o di credibile. Gli faccia prendere la parola; chieda al Governo di dare delle risposte; chieda al Presidente Conte di trovare un'altra sede, perché in questa sede non è aria per lui in questo momento,

il Governo dice che è pronto a presentare un emendamento alle ore 8 di domani mattina? Noi ci siamo, nessun rinvio per noi, si assuma la responsabilità il Governo. La ragione per cui siamo qui

l'istituzione e il lavoro del bilancio. Noi, quindi, non votiamo per riunirci domenica. Noi vogliamo andare avanti e chiediamo però, Presidente, di avere il tempo e il modo di approfondire il maxiemendamento.

Presidente, io mi permetto di fare un brevissimo *excursus* delle procedure parlamentari del passato sull'apposizione della fiducia sui maxiemendamenti alla finanziaria. Sono qui da tanti anni, ho svolto le funzioni di Capogruppo e anche di Presidente del Senato e ricordo a me stesso come alla Camera addirittura

dal Gruppo M5S).* Alla Camera dei deputati, in passato, è stata autorizzata dalla Presidenza la apposizione della questione di fiducia sui maxiemendamenti esitati dalla Commissione. Le Presidenze della Camera del passato non hanno mai autorizzato che i Governi ponessero la fiducia su maxiemendamenti non identici a quelli esitati dalla Commissione bilancio. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. Al Senato, in passato, vi è stata una maggiore elasticità, nel senso che

che conterrà argomenti che non sono minimamente passati dalla Commissione bilancio e credo che questo sia preoccupante e pericoloso. Invito i colleghi della maggioranza a prendere atto del fatto che nemmeno loro, ad oggi, conoscono il testo, perché lo sta scrivendo l'Europa,

intervengo sull'ordine dei lavori per comunicare che il nostro Gruppo, a conclusione della seduta, occuperà l'Aula per protesta contro l'atteggiamento scandaloso del Governo nei confronti del Senato.

primo Presidente donna di questa importante istituzione, mi ha intimato di stare zitta. Oggi il presidente Conte ha dichiarato che non controlla il Parlamento. Mentre chiedevo serietà lei, primo Presidente donna di questa importante istituzione, mi ha detto che

Quello che lei ha usato nei miei confronti è un linguaggio machista, appartenente a una cultura poco democratica. Vorrei ricordare, signor Presidente, che io sono una eletta dal popolo, di minoranza ma sempre eletta dal popolo. E lei, signor Presidente, non solo per il nostro Regolamento ma anche per la Costituzione che è stata conquistata anche da coloro che, come me, vengono da una cultura politica profondamente democratica e di rispetto delle minoranze,

lei che in questa sede esercito funzioni che sono date dalla Costituzione, per cui deve mettermi nelle condizioni di rispettare il mandato.

invito, quindi, proprio per il rispetto democratico che lei sta richiamando e ha richiamato più volte, a rispettare anche gli altri. Il presidente Conte stava spiegando

non mi sembrava affatto rispettoso. Così come ho ripreso lei, riprendo sempre tutti coloro che interrompono le le manifestazioni di pensiero, anche se non condivise. Questo è rispetto della dialettica parlamentare, che lei richiama continuamente ma che disattende con i fatti.

Abbiamo appreso in Aula della presenza domani del presidente Conte in Senato. Noi, quindi, ospiteremo il presidente Conte che racconterà, presumibilmente in conferenza stampa, una manovra di cui noi non conosciamo ancora il contenuto.

quello che è stato svelato dall'Europa al Governo, ma che il Governo non ha ancora svelato al Parlamento. Saremo lì, saremo presenti, lo aspetteremo e aspetteremo il suo rendiconto. *(Applausi in seduta pubblica domani, sabato 22 dicembre, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".